Presidente, vorrei sottoporre alla sua attenzione e, attraverso di lei, al presidente La Russa

e i colleghi componenti della 1a Commissione hanno, come sempre, dato il loro contributo ad un confronto non semplice, serrato, molto serio e approfondito, probabilmente sul tema più importante di questa legislatura, perché la maggioranza, con un'azione del Governo e non con un'azione parlamentare intende, proporre al Paese una modifica

abbiamo superato alcuni limiti che riguardano il rapporto non solo tra maggioranza e opposizione, ma anche tra Presidente di Commissione e componenti. Ieri al collega Magni, in un momento che probabilmente ha coinciso con una perdita di equilibrio, speriamo solo per stanchezza, del presidente Balboni, è stato detto che sarebbe stata chiamata la forza pubblica, addirittura, in una Commissione parlamentare. Devo dire di non aver mai sentito nessun collega ipotizzare l'allontanamento di un componente della Commissione con la forza pubblica: forse intendeva gli assistenti.

come proseguiamo, da qui alle prossime settimane, dentro un perimetro di regole condivise. non esiste che un Presidente di Commissione faccia valutazioni, durante una seduta, sulla natura degli emendamenti presentati dalle opposizioni. Non esiste che un Presidente di Commissione

di diritti, quelli del mio Gruppo parlamentare e quelli dei Gruppi parlamentari di opposizione. Lei non è lì per rispondere al Governo Meloni. Lei è lì per rispondere al Parlamento, al Senato. *(Applausi).* E, come lei, tutti gli altri colleghi. Glielo dico con uno spirito costruttivo, non distruttivo, perché vorrei che uscissimo da questa discussione con un accordo serio sulle regole. Sui tempi non abbiamo problemi. Possiamo passare tutto il tempo che volete, in quest'Aula e nelle Commissioni, ma i tempi devono essere decisi prima. Non esiste che si faccia un'intesa sui tempi e poi il Presidente, unilateralmente, senza nemmeno ascoltare l'Ufficio di Presidenza, decida, da un certo momento in poi, di andare avanti. Presidente Balboni, lo dico a lei, ma vale per tutti noi.

Non esiste, però, che un Presidente di Commissione decida in maniera autonoma. Non lo fa nemmeno il Presidente del Senato, pur avendone la facoltà su molti dei passaggi regolamentari. Non lo fa nemmeno il presidente del Senato, perché, anche nei momenti più critici, ci si

Nessuno di noi può dire: qui comando io e si fa come dico io, perché questa roba non appartiene alla stagione repubblicana

un quadro che rappresenta il modo in cui dovremmo provare a condurre sempre i lavori nelle Commissioni, in tutte le Commissioni e su tutti i provvedimenti. sottolineo, però, che questo provvedimento è certamente uno dei più importanti di questa legislatura, perché va a toccare parti fondamentali dell'assetto costituzionale e del nostro Stato. Va a toccare i pesi e gli equilibri tra Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio. Non posso non sottolineare come, se inizialmente la disponibilità del presidente Balboni e Balboni e dell'intera Commissione ha portato a un ciclo di audizioni completo e a una serie di interventi in discussione generale aperti a tutti i Gruppi e a tutti i membri dei Gruppi parlamentari (anch'io, pur non essendo membro

che modificano profondamente l'impianto iniziale del disegno di legge. Credo che sia corretto chiedere di tornare ad approfondire le ulteriori modifiche che il Governo - non le opposizioni - ha proposto alla Commissione e poi al Parlamento. Non riusciamo a capire il motivo della fretta su temi così delicati e importanti per il Paese intero. Non riusciamo a capire la volontà di non ascoltare le opposizioni sulle regole del gioco sulle quali poi noi ci sfidiamo democraticamente e non riusciamo nemmeno a capire il nervosismo del presidente Balboni. Forse ritiene di dover accelerare, perché magari c'è una parte della stessa maggioranza che non è così convinta di quello che si sta facendo. Non riusciamo a capire perché sull'autonomia differenziata siamo stati a discutere un periodo larghissimo, per fortuna, e su un tema così dirimente, come quello del premierato, si debba lavorare di notte, col favore delle tenebre.

ci auguriamo che ciò che è accaduto ieri sia un incidente di percorso e che si ritorni al clima necessario per affrontare il tema delle riforme di questo Paese. Noi abbiamo presentato 12 emendamenti.

cari colleghi, ovviamente non ho nessun rancore personale. Sono abituato a fare le battaglie politiche non ho paura della forza pubblica, anche perché non ho fatto niente di male. *(Applausi)*. Francamente, sono un cittadino che ha affrontato nella vita molte battaglie, anche molto più

di mettere in discussione le posizioni che noi abbiamo presentato sulla questione del premierato. Noi, a differenza dei 5 Stelle, abbiamo presentato 800 emendamenti, perché non siamo d'accordo

capacità di confronto e di discussione, in particolare con la Commissione affari costituzionali: questo è il dato. Quindi, è un problema puramente politico. Per me la questione personale è finita già ieri sera, perché le questioni personali non mi non c'entrano con la politica, però su questo punto intendo sottolineare che noi abbiamo presentato orgogliosamente 800 emendamenti perché vogliamo impedire questa riforma. Dopodiché, come ho spiegato al presidente Balboni, se fosse stato al mio posto, avrebbe fatto la stessa cosa. Quindi, in sostanza, gli ho chiesto solo di evitare questo fatto, che è stato gravissimo e inaccettabile per quanto ci riguarda.

ai colleghi dell'Assemblea che la ricostruzione offerta dal presidente Boccia è del tutto infondata. Mi dispiace, presidente Boccia, ma c'erano tanti colleghi che hanno assistito esattamente a quello che è avvenuto.

gli argomenti all'ordine del giorno erano stati stabiliti all'unanimità la settimana precedente. Tra l'altro, dei quattro punti all'ordine del giorno, due erano frutto di una richiesta delle opposizioni, alle quali avevo dato immediatamente accesso. Si era d'accordo che ieri sera si sarebbe proceduto all'inizio dell'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1, perché sull'articolo 1 non insistono subemendamenti.

tutti insieme avevamo preso quella decisione, senatore Boccia, quindi all'unanimità. Ho parlato di un'oretta, ma ne abbiamo lavorate due, e sa perché? Perché la prima ora è stata impegnata da schermaglie infinite sull'ordine dei lavori: prima si voleva rinviare la seduta, poi si volevano stabilire le regole per la settimana successiva. Ho detto al termine della seduta che avremmo svolto un Ufficio di Presidenza per stabilire come procedere nei nostri lavori la settimana successiva.

Questo è esattamente quello che è avvenuto ieri sera. È vero che ho richiamato duramente il senatore Magni; questo

stava intervenendo per illustrare i suoi emendamenti all'articolo 1; sfido chiunque a dire che non è così e ci sono i funzionari della Commissione che possiamo interpellare. Mentre la senatrice Musolino parlava, il senatore Magni si è alzato al suo fianco, incombendo su di lei e urlando a più riprese, impedendole di svolgere il suo intervento. Questo è ciò che è avvenuto. Chiamiamo i funzionari e chiediamo se è andata così o no. All'ennesimo richiamo,

è intervenuta un po' di calma, quindi li abbiamo potuti riprendere. Mi è stato rimproverato di aver alzato la voce. Ho alzato la voce, ma non sono stato né il primo, né il secondo. È chiaro che, se l'opposizione urla in Commissione, per farmi ascoltare devo urlare anch'io. Credo che questo sia fuori discussione, presidente Boccia. Forse dovrebbe spiegare al senatore Parrini che non si va sotto al banco della Presidenza a urlare e sbraitare a tutta voce; forse dovrebbe spiegare al senatore Parrini che, se ha una questione, alza la mano e chiede la parola; non viene a sbraitare a tutta voce sotto la Presidenza.

scrivete, emendando il testo del Governo, che la durata in carica del *Premier* è di un'ora, due ore o tre ore e impegnate 40 pagine di emendamenti in questo modo, mi sembra che non ci sia bisogno poi di tanto tempo per elaborare subemendamenti così complessi. Quando dico questo, senatore Magni, chi si è messo a ridere quando ha letto gli emendamenti non sono stati i colleghi di centrodestra, né il Presidente. Sono stati i senatori del PD a ridere degli emendamenti del senatore Magni. *(Applausi)*. Io non mi sono mai permesso di ridere degli emendamenti del senatore Magni; lo hanno fatto i colleghi del PD. Questa è la verità e sfido chiunque a dimostrare il contrario. Chiedo un giurì d'onore e chiedo che vengano sentiti i funzionari che erano presenti. Signor Presidente, vorrei semplicemente cercare di gettare un po' di acqua sul fuoco sulla discussione che è stata teatro delle delle questioni che sono state poste stamattina. L'invito - lo dico al Presidente - è quello di convocare un Ufficio di Presidenza *ad hoc* in cui vengano chiariti tutte queste incomprensioni, questi fraintendimenti

attento a dialogare con l'opposizione quando abbiamo affrontato il tema dell'autonomia, non vedo ragioni per cui lo stesso tipo di attenzione e di atteggiamento non possano esserci anche in occasione dell'esame di una riforma importante come quella del premierato.

tocca la Carta costituzionale e ridefinisce parti significative della nostra forma di Governo. Per rimetterla sui giusti binari, credo che però dobbiamo avere tutti chiaro

ad approfondire le loro considerazioni e ad avviare una discussione generale, che è stata anche posticipata di settimane. Al termine della discussione generale, è stato fissato un termine per la presentazione

aver bisogno di ripensare la proposta. In ogni caso, il termine - è questo che conta - era congruo e coerente con una lunghissima discussione e un lungo approfondimento. Accade poi che

è stato riscritto in gran parte, e non si dica che sono stati toccati solo alcuni aspetti, perché sono stati persino aggiunti nuovi articoli che incidono su parti prima non coinvolte, quindi anche il perimetro della riforma è stato ampliato e il contenuto ridefinito. di logica, visto che non si tratta di un decreto-legge, non c'è un termine di urgenza e stiamo parlando della Costituzione, sarebbe stato ragionevole stabilire di riconvocare gli auditi, o almeno gran parte di essi, per sentire se su questo nuovo testo fossero d'accordo o meno.

che fanno sì che ci sia il tempo necessario per convincere la maggioranza a ripensare la riforma. *(Applausi)*. Abbiamo presentato 800 emendamenti,

equilibrata, che risolve in maniera molto più efficace di quella avanzata dal Governo il tema della stabilità e del miglior funzionamento della nostra forma di Governo.

e arreca solo un danno alla nostra democrazia, speriamo di convincere la maggioranza. È la democrazia parlamentare, questa, che attraverso gli istituti che il Regolamento prevede cerca anche di prendere tutto il tempo necessario per fare breccia. Questi sono gli altri 780 emendamenti.

il Governo presenta, in sede di conversione, degli emendamenti. Abbiamo quindi ottenuto ben ventiquattr'ore per ripresentare gli emendamenti al nuovo testo come fosse un decreto-legge. Abbiamo ripresentato gli emendamenti e poi abbiamo chiesto non iniziare subito la discussione e l'illustrazione degli emendamenti, ma di prenderci il tempo per organizzare i lavori. È vero, il Presidente mi ha anticipato che intendeva iniziare la trattazione degli emendamenti relativi all'articolo 1, l'unico che non è stato toccato, perché riguarda

Allora perché iniziare l'illustrazione e quindi il percorso di una riforma costituzionale, che viene raccontata come la madre di tutte le riforme, alle ore 20 di sera, quando dalle 8,30 eravamo già in Commissione? Abbiamo detto no! *(Applausi)*. Cosa è successo? Che, a fronte della richiesta di fare una calendarizzazione dei lavori che ci consentisse di conoscere per tempo gli argomenti, ma soprattutto di conoscere per tempo quante ore dedicheremo a questa proposta,

e ragionevole di una discussione che non può essere più contratta e più mortificata di quanto avvenga quando noi convertiamo in legge i decreti-legge o di quanto è avvenuto (perché abbiamo memoria) con la discussione sull'autonomia differenziata. Signor Presidente, innanzitutto mi riallaccio all'intervento che abbiamo appena ascoltato del senatore Giorgis, che spiega anche perché, pur essendo la seduta iniziata da quaranta minuti, non siamo passati al punto all'ordine del giorno: ci ha detto chiaramente che

le loro ragioni, che hanno tutto il diritto di manifestare; ma il fatto di manifestarlo 780 volte forse è questione di misura, che è importante nelle umane cose. Dunque sono 390 ore, come abbiamo visto recentemente: un intervento per ogni Gruppo, poi ci possono essere altri interventi e altre trovate creative. Vuol dire 390 ore di lavori in Commissione, cosa che non è compatibile, evidentemente, con i lavori d'Assemblea. Ricordo che, pochi anni fa, da quella stessa parte arrivò una riforma costituzionale molto più ampia, che modificava decine di articoli della Costituzione, con sedute dalle ore 9 del mattino fino a mezzanotte inoltrata,

che, stravolgendo i lavori e ciò che è previsto dalla stessa Costituzione, ossia che si vota articolo per articolo, in un solo articolo riassumeva il contenuto dell'intera norma. Per cui di forzature ne abbiamo viste. In questo caso non abbiamo una forzatura. Abbiamo avuto dei momenti

ma la sostanza è questa: quando c'è disordine in Aula (nell'Aula dell'Assemblea plenaria, così come nelle singole Commissioni), il Presidente ha il diritto e soprattutto il dovere di mantenere l'ordine. Per cui, se stava la senatrice Musolino, aveva diritto a concludere l'intervento, così come aveva diritto il senatore Magni a parlare, ma a suo tempo. Di conseguenza, non vedo questo fatto straordinario, se non

per ogni contrasto che c'è in Commissione (e sappiamo che c'è ne sono spesso in ogni legislatura, con ogni maggioranza, con qualsiasi Presidenza), portare

il Presidente del Senato riterrà di convocare, ma io chiederei di passare all'ordine del giorno, ribadendo la correttezza del presidente Balboni, che ha un'esperienza e un'equanimità che credo gli possano riconoscere tutti. *(Applausi)*. Nei momenti di contrasto bisogna tenere presente che le reazioni sono anche proporzionate alle azioni. Di conseguenza non ci si può lamentare se il Presidente ha alzato i toni quando si è creato quello che viene definito dal Regolamento un tumulto in Aula, che era anche qualcosa più di un tumulto. Credo dunque che dovremmo chiudere qui, altrimenti dobbiamo stabilire in calendario, attraverso una Conferenza dei Capigruppo, che oggi si discute di quello che è successo nella 1a Commissione. *(Applausi)*. Martedì magari parliamo di quello che è successo nella 4a Commissione, come è già stato fatto. Direi che tutto questo non è previsto dal Regolamento e dalle prassi.

posto una questione di rispetto delle regole di civile convivenza in Commissione affari costituzionali e abbiamo chiesto alla Presidenza del Senato di adoperarsi affinché si sia certi che la Presidenza della 1a Commissione del Senato sia la Presidenza di tutti i Gruppi parlamentari e non solamente di alcuni. Abbiamo segnalato due episodi, che sono molto gravi, rispetto ai quali noi chiediamo alla Presidenza del Senato - mi rivolgo a lei, Presidente, e la ringrazio di avermi dato la parola - che ci sia la garanzia che non si ripetano mai più. Ieri in Commissione abbiamo visto infatti il Presidente della Commissione, che rappresenta tutti i Gruppi parlamentari, compiere la pratica della irrisione degli emendamenti di un Gruppo di minoranza. È una cosa che io non ho mai visto in undici anni di Parlamento. un'altra cosa che non ho mai visto in undici anni di Parlamento, Presidente, che vorrei non si ripetesse mai più e non è un problema tra me e il presidente Balboni. Come hanno fatto decine di volte, decine di colleghi, durante lo svolgimento dei lavori della Commissione, avendo io un dubbio su un'interpretazione di un punto del Regolamento, mi sono avvicinato, a a margine dei lavori, al consigliere parlamentare che in quel momento assisteva ai lavori per fargli una domanda. Non appena io ho fatto questo tutti i colleghi hanno visto che cosa è accaduto. Come se quel funzionario parlamentare fosse un dipendente del Presidente e non una persona al servizio dell'intera Commissione. Noi chiediamo che questi macroscopici abusi della funzione di Presidenza di Commissione non avvengano. Soltanto questo chiediamo. Non ci sono questioni personali.

Sono stata avvisata però di quello che è successo prima che io entrassi in Aula e so che il presidente Balboni mi ha citato. Allora, Presidente, premesso che per me la politica e l'esercizio della stessa è un'attività alta, talmente alta e qualificata, che ritengo che le polemiche e gli scontri - determinati anche dalla passione, per carità, perché ognuno di noi crede in quello che fa

a quello sfogo momentaneo. Ciò premesso, confermo che nella concitazione del momento, il presidente Balboni, dopo aver ascoltato la nostra richiesta, come forze di opposizione, di non procedere alla discussione degli emendamenti, avendo bisogno di più tempo per poterli illustrare,

esercitando ovviamente il suo ruolo di Presidente. A quel punto il primo emendamento era quello di Italia Viva, a firma mia e del senatore Borghi, quindi toccava a me iniziare la discussione, ma gli animi erano talmente accesi che in sostanza i colleghi continuavano a parlare e quindi io non riuscivo a svolgere il mio intervento. Questo si è ripetuto per due volte. Da qui in poi il presidente Balboni ovviamente è intervenuto in maniera ancora più vigorosa per ristabilire la correttezza per ristabilire la correttezza dello svolgimento dei lavori e anche un po' di tranquillità. In seguito - proprio per dare una cronaca dei fatti - ho chiesto al Presidente di avere una breve sospensione, funzionale più che altro a cercare di riportare un po' di tranquillità e di serenità negli animi di tutti i commissari presenti; la sospensione è stata immediatamente accordata dal Presidente, abbiamo sospeso cinque minuti e poi ho svolto il mio intervento. Questi sono i fatti.

che riguarda in realtà un tema abbastanza rilevante. Con l'articolo 2 del disegno di legge Nordio si interviene sul codice di procedura penale con alcune previsioni che, in sé, introducono principi con i quali noi non siamo in contrasto. Riteniamo, cioè, che si tratti di principi anche condivisibili. Tuttavia, pensiamo che

da parte della maggioranza, anche rispetto alle nostre posizioni. Questo ascolto non c'è stato e, se posso permettermi, mi rammarico molto che, durante la discussione in Commissione, poi durante la discussione generale in Aula e anche adesso durante il voto degli emendamenti, il ministro Nordio non abbia mai sentito la necessità di essere presente, in Aula o in Commissione,

sia importante, sia rilevante. Forse, ritiene anche lui che si tratti di un provvedimento che non porterà di fatto alcun beneficio e che non avrà alcun impatto sulla nostra giustizia. In tal caso si capirebbe perché preferisce non metterci troppo la faccia. sull'emendamento in particolare, che riguarda l'interrogatorio di garanzia, noi siamo in linea di principio favorevoli a un interrogatorio di garanzia che preceda l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. È un principio corretto, che però deve essere declinato nel modo giusto. Bisogna evitare, cioè, che l'interrogatorio di garanzia diventi un grimaldello attraverso il quale la misura risulti impossibile perché previene la possibilità di una sua applicazione. Noi abbiamo proposto una serie di emendamenti, anche sulla scorta delle indicazioni che ci sono venute da autorevoli figure, come il procuratore nazionale antimafia, il dottor Melillo, che suggeriva di escludere dall'applicazione di questa norma almeno alcune fattispecie di reato, sulle quali interverrà in particolare la collega Rando. Non vi è stata, però, alcuna apertura neanche a queste modifiche. Rimane, quindi, una norma che introduce un principio corretto, che tuttavia noi riteniamo potesse essere declinato meglio. anche perché l'impatto che avrà questa misura sul piano concreto sarà molto limitato, perché, come è possibile leggere nel provvedimento, si tratta di una misura che non si applicherà quando la misura cautelare della custodia in carcere debba essere applicata in ragione del pericolo di fuga o del rischio di inquinamento delle prove, cioè per i due motivi che, nella stragrande maggioranza dei casi, vengono utilizzati per chiedere la custodia cautelare. Verrà utilizzata solo per l'ipotesi di rischio di reiterazione dei reati, quindi solo in casi residuali. Quindi, il nostro voto favorevole a questo emendamento soppressivo dipende soprattutto dal modo in cui è stato realizzato questo intervento, non tanto dal principio in sé.

perché prevede la possibilità di parlare di interrogatorio preventivo anche per i delitti che concernono il codice rosso. Allora, noi in quest'Aula e nelle Commissioni di pertinenza abbiamo lavorato tantissimo al codice rosso, siamo arrivati a un assetto normativo di tutto rispetto abbiamo fondato il nostro lavoro sull'intento di accelerare la tutela delle donne e di svolgere un'attività preventiva della violenza sulle donne. Ora, ammettere un interrogatorio preventivo è contro tutta la *ratio*

Signora Presidente, vorrei solo ricordare alla senatrice Lopreiato che l'emendamento 2.134 non ha nulla a che vedere con il codice rosso, ma semplicemente prevede di restringere ai reati di criminalità organizzata, per i quali può non essere disposto l'interrogatorio preventivo con riferimento alla custodia cautelare richiesta per il pericolo di reiterazione del reato. Quindi, non ha nulla a che vedere col codice rosso, ma riguarda un'altra tipologia di reato. *(Applausi)*.

prevede una riforma dell'articolo 291 del codice di procedura penale, che introduce un trattamento privilegiato nella procedura di applicazione delle ordinanze di custodia cautelare per i reati tipici dei colletti bianchi. Attualmente, le ordinanze di custodia cautelare possono essere emesse ed eseguite immediatamente, anche nei casi nei quali sussiste il concreto e attuale pericolo che l'indagato, se viene lasciato in libertà, commetta altri delitti della stessa specie di quello per cui si procede. La riforma in esame prevede che la normativa vigente resti in vigore per i reati commessi con violenza, per reati in ambito di criminalità organizzata, per reati in codice rosso contro le fasce deboli, per reati con uso di armi, per reato di maltrattamento in famiglia, per reato di contrabbando di tabacchi esteri, per reati di associazione a delinquere semplici. Tenuto conto che, guardando la casistica nazionale, si tratta della quasi generalità dei casi per i quali vengono attualmente emesse le ordinanze di custodia cautelare, la domanda è: ma allora qual è la novità introdotta con il disegno di legge in esame? La novità è che, mediante una chirurgica modifica dell'articolo 291, è stato creato un trattamento differenziato privilegiato, riservato a una ristretta categoria di indagati, cioè gli indagati per i delitti commessi senza violenza, ossia tipicamente quelli propri dei colletti bianchi: gli atti di corruzione, di riciclaggio, illeciti finanziari, reati di bancarotta ed altri. Per questa categoria di reati, grazie a questa riforma, l'ordinanza di custodia cautelare non potrà più essere eseguita subito se sussiste il rischio di reiterazione di reati della stessa specie; dovrà essere sospesa e notificata all'indagato almeno cinque giorni prima della sua esecuzione, con il contemporaneo deposito in cancelleria di tutti gli atti di indagine. Solo dopo questo adempimento, il giudice potrà procedere all'interrogatorio dell'indagato, sempre in stato di libertà. Ma se l'indagato deve essere avvisato in anticipo che è stata richiesta una misura cautelare nei suoi confronti e per di più deve essere effettuata la *discovery* anticipata di tutti gli atti di indagine compiuta, è evidente che si crea con ciò stesso il pericolo - magari prima inesistente - che l'indagato si dia alla fuga o che egli o i suoi complici ancora non individuati e per i quali le indagini sono in corso facciano sparire il bottino o documenti essenziali, oppure intimidiscano e corrompano i testimoni. Per questa ragione abbiamo proposto un emendamento che preveda che l'attuale regime sia previsto anche per i reati più gravi di corruzione e che quindi l'ordinanza sia eseguita e che dopo si proceda all'interrogatorio. Non capiamo perché si debba mantenere questo regime per reati di contrabbando di sigarette, perché si debba mantenere per associazione a delinquere e non si debba mantenere per corruzione per milioni di euro. Se così è, questa è l'ulteriore declinazione del fatto che, dietro tecnicismi incomprensibili per l'uomo comune, si nasconde una concezione classista del diritto penale.

per un messaggio preciso alla lotta alla criminalità organizzata. Che cosa prevede questo emendamento dicendolo in maniera chiara? L'interrogatorio è sempre escluso nei casi in cui si procede per delitti gravi. Stiamo parlando di riciclaggio, di atti di violenza con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, di reati commessi con metodo mafioso o con agevolazione dell'attività

Vorrei ricordare non soltanto ai colleghi, ma magari a chi segue anche il dibattito, cioè ai cittadini, che stiamo parlando di un intervento che potrà eventualmente realizzarsi già per disposizione contenuta in questo provvedimento soltanto tra oltre due anni, perché potrà realizzarsi soltanto se e quando entreranno nelle piante organiche ben 250 magistrati in più.

l'entrata in vigore di un collegio, con ben tre giudici impegnati su questo punto della custodia cautelare, creerà tra l'altro una serie di incompatibilità,

del sistema. Nella mia Regione, per esempio, il tribunale di Ivrea lancia segnali di grande allarme e disperazione, perché deve affrontare inchieste molto importanti, da ultima

Addirittura - credo anche un po' provocatoriamente - all'inaugurazione dell'anno giudiziario qualcuno ha proposto di tornare indietro rispetto alle circoscrizioni giudiziarie, togliendo loro parte delle competenze, che è obiettivamente peggio che uscire con le mani alzate.

su cui - come sappiamo - si è già intervenuti ripetutamente con interventi legislativi negli anni scorsi. Sappiamo che è in discussione alla Camera una ulteriore proposta di modifica della prescrizione, che punta a ripristinare il vecchio regime della prescrizione sostanziale. Noi riteniamo che sia quella proposta, sia questa, che mirano entrambe a superare l'assetto definito e delineato dalla riforma

per il fatto, semplice ma ineludibile, che la riforma Cartabia ha introdotto un principio per noi molto interessante, molto innovativo, e cioè quello della prescrizione processuale, ossia che, se se i processi in appello non vengono celebrati entro un certo termine, si debbono concludere e perdono di efficacia. Quel principio è stato molto innovativo per il nostro sistema giudiziario;

direi clamorosi sulla durata dei processi di appello in Italia, che sono il vero tallone d'Achille del nostro sistema processuale penale. Sappiamo che la durata dei processi penali in Italia è molto, molto superiore a quella media dei processi nel resto d'Europa, soprattutto per la durata eccessiva dei processi d'appello. Per effetto dell'introduzione della prescrizione processuale, cioè della riforma Cartabia, che sia questa proposta emendativa del senatore Scarpinato, sia quella che è in corso di discussione alla Camera vogliono superare, superare, i tempi dei processi in appello, soprattutto nei distretti di corte d'appello dove duravano in maniera inaccettabile, in un anno e mezzo si sono dimezzati. Abbiamo le statistiche del Ministero della giustizia. Per esempio, nel distretto della corte d'appello di Napoli nel giro di un anno e mezzo, la durata dei processi è passata da oltre duemila giorni a meno di mille giorni. Questo perché quel principio introduce una forma di responsabilizzazione dei dirigenti degli uffici giudiziari, che evidentemente li induce a una maggiore organizzazione dell'ufficio giudiziario, in grado di garantire una tempistica più adeguata e più coerente con le necessità della giustizia. Per noi tornare indietro da quell'assetto senza prima averne verificato e misurato in concreto gli effetti, che già oggi appaiono molto confortanti, è un errore, tanto più in un momento in cui la durata dei processi è il criterio principale su cui l'Europa misura l'efficienza e la capacità di riforme del nostro Paese in vista dell'erogazione dei fondi del PNRR. Pertanto, tutte le ipotesi come quella in puntano a superare quella riforma, secondo noi in questo momento sono sbagliate. comprendo le motivazioni che sono state svolte dal senatore Bazoli. Tuttavia, vorrei ricordare che, in occasione dell'inaugurazione dell'ultimo anno giudiziario, il presidente della corte d'appello ha detto che sono pendenti dinanzi Ci sono decine e migliaia di procedimenti pendenti presso la corte d'Appello di Napoli, che non potranno essere definiti nei tempi previsti dalla Cartabia. E allora avremo una falcidia di questi procedimenti perché, non adeguando il numero dei magistrati al numero dei processi, saranno destinati alla improcedibilità. Ecco perché noi abbiamo insistito per questo emendamento.

e importante. Esso riguarda la previsione della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte dei pubblici ministeri.

per la pubblica accusa di contestare una decisione del tribunale che riconosce l'innocenza di una persona al termine del processo di primo grado. Si tratta di un principio sul quale è giusto discutere è giusto discutere perché, mentre i principi di diritto anche sovranazionali riconoscono come un principio ineludibile fondamentale il riconoscimento dell'imputato che sia stato condannato

non altrettanto può dirsi per un diritto della pubblica accusa ad impugnare una sentenza di assoluzione perché questo non è coperto dallo stesso principio. Ovviamente uno Stato, che ha avuto la possibilità di indagare con i poteri soverchianti che sappiamo essere appannaggio della pubblica accusa durante le indagini preliminari nei confronti di ciascun singolo cittadino, cittadino, non sia stato poi in grado di dimostrare la colpevolezza della persona dopo il processo di primo grado,

tentare di dimostrare la colpevolezza della persona indagata, pur dopo esattamente che un tribunale abbia già detto che quella colpevolezza non c'è.

Questa strada venne appunto tentata con la famosa legge Pecorella, con la quale si pensò di introdurre questo principio; questo principio; ma quella norma, introdotta con la legge Pecorella, venne dichiarata incostituzionale dalla Corte, sulla base di alcune considerazioni che noi riteniamo, almeno in parte, non superate da questa nuova proposta. Questa nuova proposta, rispetto alla legge Pecorella, introduce una distinzione, cui l'inappellabilità varrebbe solo per alcune categorie di reati meno gravi e non per quelli più gravi. che affrontava il tema in maniera secondo me più intelligente - posso dirla così? - più ragionevole e più equilibrata di quanto sia stato fatto in questo disegno di legge. Era la proposta della Commissione Lattanzi, sulla quale abbiamo provato a a innescare una discussione in Commissione, purtroppo senza successo per la rigidità che c'è stata sempre su questo provvedimento da parte della maggioranza. Quella proposta introduceva il principio dell'inappellabilità del pubblico ministero, ma lo faceva dentro una cornice di riforma dell'impugnazione e dell'appello, che la rendeva - secondo noi - molto più equilibrata e soprattutto non soggetta ai rischi di incostituzionalità che questa norma invece si porterà dietro. Secondo noi quella era la strada da intraprendere.

che le impugnazioni dei pubblici ministeri avverso le sentenze di proscioglimento sono l'1,4 per cento del totale delle impugnazioni. Quindi, l'effetto deflattivo che avrà questa riforma è poco più di zero, tanto per essere chiari. Stiamo parlando di una cosa che ha un effetto molto limitato e che si presta ancora a obiezioni di costituzionalità. Si poteva fare molto meglio.

Intanto, è contraria a ogni elementare senso comune. È in contrasto con qualsiasi senso comune ritenere che il giudice di primo grado possa commettere degli errori quando condanna l'imputato e non sbagli mai quando invece assolva l'imputato. Il senatore Zanettin, relatore di maggioranza, per ridimensionare la portata di questa riforma, ha detto che tutto sommato riguarda soltanto reati minori, come quelli previsti dall'articolo 550 del codice procedura penale con citazione diretta. Mi meraviglia questa affermazione del senatore Zanettin. Il senatore Zanettin sa benissimo che non è vero. L'articolo 550 prevede reati che sono puniti sino a dieci anni di galera: il furto pluriaggravato è punito fino a dieci anni; le lesioni personali gravi o gravissime per incidente stradale sono punite sino a sette anni; la ricettazione è punita sino a otto anni. Come si fa a dire che sono reati minori? Questo determina una gravissima lesione del diritto delle vittime. Abolito il potere del pubblico ministero di appellare e siccome alle vittime non è dato il diritto di appellare, si realizza una grave ingiustizia. Mi meraviglio di Fratelli d'Italia, che - da una parte - propone di introdurre una riforma della Costituzione per garantire i diritti alle vittime e - dall'altra - calpesta, con questa riforma, i diritti delle vittime. Il senatore Zanettin, consapevole che questa tipologia di riforma è stata già bocciata dalla Corte costituzionale nel 2007, per contrasto con l'articolo 111, invece di contro argomentare giuridicamente rispetto alle motivazioni di quella sentenza, ha usato la facile scorciatoia della delegittimazione della Corte costituzionale, affermando che quella sentenza era motivata dal furore ideologico anti-berlusconiano e replicando l'accusa di Berlusconi alla Corte costituzionale di essere un covo di comunisti. Questo è il senso delle istituzioni che ha questa maggioranza. La Corte dichiarò l'incostituzionalità argomentando il contrasto con l'articolo 111, perché affermò che la simmetria tra i poteri del pubblico ministero e quelli dell'imputato, vietando si giustifica solo se vi siano ragioni di economia processuale e se c'è un interesse generale. Così si limita il potere di appello del pubblico ministero in certi casi di giudizio abbreviato, come come contropartita al fatto che l'imputato, col giudizio abbreviato, rinuncia al contraddittorio del dibattimento. Così si vieta il potere di appello del pubblico ministero per le condanne e per tutti i reati previsti con l'ammenda, perché così si deflaziona il carico dei processi penali. Ma qual qual è la contropartita per lo Stato, che riequilibra le posizioni tra le parti con un divieto d'appello per reati fino a dieci anni? Quindi, questa norma è assolutamente irragionevole.

il collega Bazoli - l'estrema preponderanza di mezzi che l'accusa ha sulla difesa, chi potrà mai dire che la condanna in appello sia stata oltre ogni ragionevole dubbio? Se non è un dubbio sulla colpevolezza una sentenza di proscioglimento in primo grado, vi chiedo - care colleghe e cari colleghi - che cosa è più dubbio di quello? Se una corte della Repubblica, in nome del popolo italiano ti ha mandato assolto, vuol dire che il dubbio sulla tua colpevolezza permarrà sempre. Noi abbiamo avuto in questo paese persone, come paese persone, come Adriano Sofri, che è stato condannato, per un reato molto grave, dopo aver visto sentenze suicide, sentenze scritte dal relatore in modo contraddittorio al dispositivo,

Vero, senatore Scarpinato, ma il prezzo dell'errore del giudice di primo grado non lo deve mica pagare l'imputato. *(Applausi)*. Io chiedo al senatore Scarpinato che sanzione c'è? In quale sanzione incorre il magistrato di primo grado che ha preso una decisione di assoluzione sbagliata? Se vogliamo tutelare le vittime del reato, non lo si fa caricando il peso dell'inefficienza della giustizia sul povero cittadino che, assolto in primo grado, non è libero di tornare alla sua vita civile, perché deve affrontare un secondo grado. E questo perché, come dice il collega Scarpinato, i giudici sbagliano in un senso o in un altro. Allora, se il giudice sbaglia, che ci sia una sanzione per il giudice che sbaglia in modo marchiano. In Commissione si è fatto un caso concreto. Io voglio rivolgermi alla collega Cucchi, che ha condotto una battaglia civile non solo per se stessa, ma per tutto il popolo italiano, nel difendere la sua causa. Quello che dico è che la sentenza di primo grado, che ci indignò, che ci indignò, vide i magistrati che la emisero uscire completamente indenni da quell'indignazione di tutta l'opinione pubblica. Allora davvero vi dico: non ci fermiamo davanti alla giurisprudenza della Corte costituzionale, perché -

davanti a nuovi ritorni del legislatore, modificarsi. Lo abbiamo visto già più di una volta: le sentenze delle Corti supreme non sono scritte nel marmo e non cambiano più. Allora vi sfido, cari colleghi e cari colleghi, a trovare una fallacia logica in quello che dico. Ribadisco: penso che, se un cittadino è dichiarato innocente da un tribunale della Repubblica, debba poter tornare alla sua vita e non sottostare a una spada di Damocle che gli viene posta per l'errore del magistrato. È inaccettabile.

Signor Presidente, noi sappiamo bene che l'intento del legislatore è trovare quelli che sono *escamotage* per snellire i carichi giudiziari. Lo fa anche in sede civile, anche se purtroppo noi della giustizia civile ne parliamo poco in Commissione - parlo, ad esempio, della mediazione, oppure della negoziazione assistita

noi con l'emendamento 2.162 ripristiniamo l'esclusione del concordato preventivo di appello su determinati reati, proprio per la gravità degli stessi; in particolar modo parliamo dei delitti di mafia e terrorismo e dei reati sessuali, dove

capito - lo dico con pacatezza - si tratta del monitoraggio dei dati conseguente alla riforma Cartabia, con particolare riferimento alla questione

pensiamo che il monitoraggio previsto dalla riforma Cartabia, alla quale abbiamo tutti contribuito, fosse proprio la misura di quell'approccio che dovremmo tutti avere a tutte le leggi che approviamo, ma soprattutto quando introduciamo delle innovazioni sul sistema giustizia. Occorre cioè innanzitutto monitorare, raccogliere i dati e intervenire laddove e se necessario. Anche per questo

a provocare la paralisi, perché sappiamo che tra poco arriverà l'ennesima modifica in tema di prescrizione, che creerà di nuovo dei problemi; c'è sempre da intervenire su quello che è stato

si era quando c'erano i problemi. Quando c'erano i problemi, il Partito Democratico non solo c'era, ma ha fatto anche proposte accoglibili, che sono state accolte e hanno avuto un loro effetto. e hanno avuto un loro effetto. Visto che si è parlato molto di custodia cautelare, vorrei ricordare che nel 2015 il Partito Democratico ha proposto e ha fatto approvare una modifica maggiori garanzie sul pericolo di reiterazione del reato proprio sulla custodia cautelare, intervenendo non per escluderla e fare un liberi tutti indiscriminatamente, ma sull'aspetto cruciale della motivazione, che può ovviamente essere migliorato. Ricordo a me stessa e all'Assemblea che il partito della Lega votò convintamente contro, paventando che ci sarebbero stati eserciti di delinquenti in giro per le strade e che avremmo messo tutti fuori: questo a proposito di chi si proclama garantista nella fase delle indagini preliminari e molto giustizialista nella fase dell'esecuzione.

lo smaltimento dei processi. Per questo la proposta ha un'efficacia limitata al 31 dicembre 2026, ovverosia alla previsione dello svolgimento di quei concorsi volti a sopperire alla carenza di personale. Allo stesso tempo prevede che i magistrati che vogliano rimanere in servizio possano essere collocati d'ufficio nei settori più critici con riferimento alle pendenze, alla scopertura degli organici e sempre e comunque all'interno del medesimo circondario. Nel contempo viene mantenuta a settant'anni la decadenza dagli incarichi direttivi, al fine di consentire gli avvicendamenti già previsti e fisiologici nel governo interno della magistratura.

vorrei fare presente che il tema è stato oggetto di una serie di approfondimenti, ma c'è il parere contrario da parte della 5a Commissione. Quindi su questo testo il parere contrario è legato proprio al tema economico.

Già in passato c'erano state ipotesi di mantenimento in servizio di magistrati; tutte ipotesi che poi non hanno trovato compimento - secondo me

del giudizio collegiale per convalidare una misura cautelare sarà tra due anni, in attesa di nuovi ingressi di magistrati. Ieri il nostro capogruppo in Commissione giustizia Bazoli diceva che non lo applicherete mai, perché è evidente che c'è un cronico ritardo sia nell'arretrato, nello smaltimento del pregresso (nonostante i risultati che già le riforme Cartabia hanno prodotto), sia nella lentezza delle procedure per l'assunzione di nuovi magistrati.

vi sbrighiate a trovare modi corretti e sostenibili costituzionalmente per accelerare l'ingresso di magistrati in servizio, così da poter svolgere i loro compiti per una durata ragionevole dei processi, oppure si prendano in considerazione altre forme.

il mantenimento in servizio di magistrati specialmente in alcune aree e in alcuni uffici giudiziari dove la mancanza avvenisse senza il mantenimento di incarichi direttivi da parte degli stessi magistrati, ma magari al servizio dei momenti collegiali di giudizio o di altre attività degli uffici giudiziari, potrebbe essere una sorta di

che l'emendamento, che non voteremo, pone un problema e il Governo deve aiutare a risolverlo o con l'accelerazione dell'entrata in servizio di nuovi magistrati, quelli che servono, oppure prendendo in considerazione,

non sono riuscito a votare, nonostante la sua cortesia, l'articolo 2. Detto questo, rilevo ancora che disturbo, in questo luogo troppo stretto, sia non potendo far passare agevolmente i colleghi e le colleghe senatrici,

Senatore Guidi, le dico che averla in quest'Aula per noi è una ricchezza e un dono. Quindi, faremo di tutto per far sì che lei sia sempre più a suo agio.

partendo da un dato di realtà. Sappiamo che mancano circa 1.500 magistrati. Abbiamo sentito, in occasione dell'inaugurazione dell'ultimo anno giudiziario, l'esposizione di situazioni incredibili. Alla procura di Ivrea hanno l'80 per cento dell'organico in meno e hanno intercettato delle conversazioni di criminali che proponevano di andare lì a commettere reati perché tanto non sarebbero mai arrivati a processarli. È un dato processuale. Sappiamo che con i concorsi i nuovi magistrati prenderanno servizio tra due o tre anni, ma nel frattempo, per il naturale *turnover* a seguito dei pensionamenti, si verificheranno dei vuoti di centinaia di altri magistrati. Come dobbiamo fare, allora, per far funzionare questa giustizia? Ci sono delle proposte che sono assolutamente incostituzionali, come quella di assumere i giudici onorari con concorsi semplificati, dequalificando il livello di preparazione della magistratura. Diventa invece razionale che, se abbiamo dei magistrati che hanno una grandissima esperienza di carriera,

teniamo in piedi la baracca, cercando di non far crollare il sistema, Non si può dire che la giustizia non funziona per un destino cinico e baro: non funziona perché questa maggioranza non sa prendere le decisioni che qualsiasi padre di famiglia prenderebbe.

In Commissione giustizia abbiamo sentito gli esperti, tra cui alcuni che hanno ricoperto ruoli dirigenziali al Ministero della giustizia, i quali ci hanno spiegato quanto segue. In Italia ci sono più di cento piccoli tribunali, che hanno un organico tra i 18 e i 21 magistrati. Se si introduce il giudizio collegiale, i magistrati che faranno parte del collegio diventeranno automaticamente incompatibili per tutti i giudizi penali nei confronti degli stessi imputati, per tutti i provvedimenti a carattere di intercettazione e per i giudizi abbreviati: si determinerà la paralisi. Abbiamo fatto quindi il conto della serva.

Non è che la paralisi si verifica all'improvviso, ma perché questa maggioranza vuole fare le nozze con i fichi secchi. Non si possono fare giudizi collegiali, se non si aumentano i magistrati. Abbiamo quindi proposto

5 cercano di fare una cosa che questo provvedimento non fa, cioè di intervenire per migliorare il servizio e l'efficienza della giustizia nel nostro Paese. Sono tutti emendamenti aggiuntivi, che, certo, impegnano risorse, perché sappiamo che per per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi della giustizia bisogna spendere qualche soldo. Non casualmente, sono tutti emendamenti sui quali c'è il parere negativo.

senza però premurarsi di spiegare come questo sarà possibile, dato che, come ci ha detto tutti i magistrati che abbiamo audito, in questa condizione, con questo numero di giudici, la misura è di fatto impossibile. Non ci sono cioè abbastanza giudici per fare il collegio per le misure cautelari. Questo provvedimento prevede un aumento dell'organico di 250 unità; per carità, meglio di niente, ma a fronte di una scopertura attuale degli organici della magistratura che

Come sempre però, soprattutto quando si parla di giustizia, bisogna bilanciare le scelte che si fanno con le risorse disponibili. Altrimenti infatti si lanciano grandi proclami che poi rimangono sulla carta e non verranno mai realizzati, come succederà in questo caso, tant'è vero che avete previsto che

Certamente tra due anni l'organico della magistratura non sarà stato colmato per consentire di avviare una misura di questo genere.

Il fatto che esprimiate invece un parere negativo dipende ovviamente dalla scelta politica di non mettere risorse sulla giustizia. Ricordo sotto questo profilo che nel bilancio pluriennale dello Stato

proposta di legge, che però evidentemente non sarà in grado di mantenere.

Siamo molto convinti dell'idea che per privare qualcuno della libertà personale ci sia bisogno del giudizio di tre magistrati. Di conseguenza, chiediamo di assumerne di più; fosse stato per noi, la norma sarebbe entrata in vigore subito. Devo dire infatti che mi lascia un po' perplesso la carenza di logica delle votazioni come le andremo a vedere. che infatti propongono l'udienza collegiale non voglio assumere i magistrati, coloro che invece per due giorni ci hanno detto e hanno votato contro l'udienza collegiale, chiedono nuovi magistrati. Viene da chiedersi a quale fine, collega Scarpinato, sempre per il tramite della Presidenza, lei chiede 500 nuovi magistrati quando ci ha detto in tutti i modi di essere contrario a questa innovazione. Dato che invece noi siamo favorevoli, vorremmo attrezzare questa riforma con gli strumenti necessari e, di conseguenza, voteremo favorevolmente a questo emendamento e credo, più o meno, a quasi tutti gli altri riferiti all'articolo 5, perché genuinamente desideriamo che la riforma abbia anche le ruote per camminare. sia un caso più unico che raro - esprimeremo un voto favorevole all'emendamento Scarpinato, perché abbiamo fortemente sostenuto e voluto che l'applicazione delle misure cautelari sia in capo non a un giudice monocratico, ma a un giudice collegiale.

Il Governo potrebbe anche considerarne non 500, ma un numero diverso; certo però la necessità di aumentare il numero dei magistrati è un'esigenza consequenziale all'approvazione di questa riforma.

che non ci pare assolutamente anticostituzionale, perché si entrerebbe comunque per concorso, ossia di riconoscere le professionalità degli operatori del diritto che abbiano maturato un'esperienza talmente importante da consentire loro di fare un concorso semplificato. Mi riferisco ai professori ordinari di materie giuridiche nelle università e agli avvocati con più di vent'anni di esperienza. A questi professionisti, che appunto abbiano tale particolare tipo di maturità e di conoscenze, potrebbe essere richiesto di fare un concorso (quindi sempre una procedura selettiva), ma soltanto con uno scritto e un orale, con l'annotazione, molto importante, che questi nuovi magistrati, così reclutati, sarebbero addetti esclusivamente alle materie concernenti l'oggetto del concorso. Ad esempio, se parliamo di un avvocato civilista, che farà lo scritto e l'orale

innovativa, se volete, tesa però a riconoscere professionalità che già esistono a livelli molto alti. È una procedura assolutamente selettiva, che adibisce il vincitore di concorso soltanto alla materia nella quale quelle conoscenze sono state maturate. Come ho detto, non mi pare ci sia nessun problema di carattere costituzionale, né come ha detto qualcuno durante il dibattito in Commissione - si andrebbe ad abbassare il livello qualitativo della nostra magistratura. Non si pensi infatti che un professore di materie giuridiche all'università o un avvocato, che abbia per così tanto tempo esercitato la professione e superato un concorso, siano

sia necessariamente più qualificata di qualcuno che fa il professore universitario e che comunque ha fatto il concorso su quella materia; non penso proprio che questo problema si ponga. Se volete, è una maniera creativa, ma comunque efficace, anche senza dover estendere oltre i limiti della ragionevolezza l'età della quiescenza. Tra le altre cose, ovviamente, nel momento in cui cui pensassimo di estendere l'età per andare in pensione per una categoria professionale, è ovvio che il fenomeno dell'emulazione si creerebbe anche per altre professionalità, di cui pure la Repubblica ha bisogno. Penso, per esempio, ai medici e al personale sanitario. Quindi, piuttosto che ricorrere all'estensione dell'età per il trattamento di quiescenza, pensiamo che far leva su professionalità già esistenti in una modalità come quella di cui si parla in questo emendamento possa essere una soluzione.

numerica, ma di sostanza e differenza di impostazione. Noi pensiamo, infatti, che nel palazzo della giustizia la circolarità e la ricchezza delle esperienze siano esattamente ciò che manca: non una rigorosa separazione e ghettizzazione delle esperienze, come invece ci si prepara a fare in un altro ramo del Parlamento. Proprio a garanzia di una cultura plurale, in cui il contraddittorio entri anche nel procedimento di esame e intellettuale, pensiamo che debba essere innanzitutto applicato e poi sviluppato l'articolo 106 della Costituzione, che prevede che l'avvocatura possa, a certe condizioni, contribuire a esercitare la giurisdizione. Da questo punto di vista, serve un intervento legislativo. Sarebbe un intervento e un ragionamento attuale e moderno, dopo che abbiamo ormai già scolpito nella pietra e attuato il fatto che, in pratica, non si può più passare dalla funzione requirente a quella giudicante. Proprio per evitare una serie di irrigidimenti e di autoreferenzialità, la ricetta più giusta è aprire le porte, nella circolarità delle esperienze, ed evitare una cultura autoreferenziale. Con questo spirito abbiamo anche

votare questo emendamento, perché la questione è molto più pregnante e più seria di così. Da questo punto di vista, vi sarà ovviamente una nostra proposta di legge,

quello di una *task* *force* che interviene per supportare gli uffici, ma ha e avrebbe un'ambizione maggiore, cioè quella di inserire

competenze che sarebbero molto utili nei nostri tribunali: ad esempio, quando si discute di diritto fallimentare, sarebbe molto utile avere competenze di arricchimento e di supporto specifico su alcune questioni economiche, in particolar modo quando si affrontano grandi processi che hanno questo tipo di profilo, oppure nelle questioni organizzative. Insomma, per tutti quegli approfondimenti, nell'ottica che ormai conosciamo, quale si lavora sempre di più in un lavoro di squadra e di supporto, sarebbero le strade nuove che il nostro sistema della giustizia, che è al servizio dei cittadini, ha bisogno di percorrere. avevamo usufruito anche dei fondi del PNRR per introdurre questi addetti all'ufficio del processo. Tra l'altro, noi l'avevamo molto supportato, perché ha fatto sì che potessero fare ingresso in un mondo del lavoro intellettualmente specializzato e qualificato anche molti giovani. La richiesta di questo emendamento è di stabilizzare questi addetti all'ufficio del processo con contratti a tempo indeterminato, una parola che ci pare ci pare desti qualche fastidio nella maggioranza; lo vediamo anche quando discutiamo di altri provvedimenti o quando parliamo di un'occupazione che sarebbe incrementata. Peccato che ci si dimentichi di dire che è un'occupazione perlopiù precaria e sappiamo che cosa voglia dire occupazione occupazione precaria. Allora, qui c'è un'occasione: qualche sforzo sicuramente è stato fatto, ma,

vi è un controsenso: per la prima volta nella storia, grazie al PNRR e ad alcuni fondi che erano stati stanziati precedentemente, la giustizia vedeva

virgola" per la giustizia. Qua entravano quasi 3 miliardi nel comparto giustizia. Si dà il caso, però, che questa maggioranza abbia previsto una riduzione del 10 per cento in tre anni e dire che si vorrebbe fare, ma non si può è esattamente dire che non siamo, come ci viene spiegato spesso, una maggioranza e un Governo finalmente politici. Infatti, se non è politica la scelta di quali fondi e quali spese privilegiare, anche nelle politiche fiscali - e qui un bel tacer non fu mai scritto, come si suol dire mi chiedo dove sia la politica. Se non si devono trovare per queste priorità i soldi e non per altre, mi chiedo dove sia il primato della politica. In questo caso, come in altri casi, ci raccontate cose che non esistono e vi vantate di cose di cui non avete assolutamente né il dominio, né la padronanza, ma - ahimè - per scelta e non per sorte.

dopo due giorni di discussione sulla sua riforma, rispetto alla quale sono intervenuti non solo membri della Commissione giustizia, quindi sarebbe interessante anche ascoltarli.

in maniera totale alla giustizia minorile italiana. Lei lo sa meglio di me, signor Ministro, perché è espertissimo in questo campo: la giustizia minorile italiana è stata per anni un modello a cui l'Europa ha guardato con ammirazione, perché perché abbracciava il paradigma educativo, dicendo che il ragazzo può essere accompagnato e che, a fianco al fatto di dover

La giustizia penale minorile in Italia infatti non si basa - fortunatamente, diciamo noi - solo sulla valutazione del fatto, ma anche sulla persona del minore e tiene conto quindi anche della fragile transizione adolescenziale che è già difficile di per sé e che, se viene svolta in un contesto di ulteriore fragilità, mette in seria difficoltà tutto il percorso di recupero del minore. La bellezza dell'ordinamento italiano è data anche dal fatto che c'è una vera sinergia anche con i principi internazionali che sono stati condivisi con l'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989. Non è un approccio buonista quello di dire che si deve mettere al centro il minore con le sue fragilità e capire quali possano essere le strategie di recupero, quindi non pensando solo alla pena, ma per fare questo abbiamo bisogno di figure

Il carcere per quei ragazzi è sempre un'esperienza traumatica, che rischia di cristallizzare in senso negativo l'identità fragile del minore, proprio nel periodo più delicato di quel passaggio adolescenziale. Avremmo quindi bisogno di potenziare le comunità di accoglienza,

Ministro, a questa emergenza sociale ne associo un'altra, perché queste figure educative mancano anche per un altro aspetto. Signor Ministro, lei sa, ma non è colpa sua - vedo anche il Ministro per la pubblica amministrazione, abbiamo bisogno di fare un lavoro tutti

facendo le notti e i turni. Abbiamo bisogno di lavorare anche per dare dignità a questo mestiere, perché, se pensiamo che l'educazione sia al centro, allora va valutata anche nel riconoscimento sociale di chi svolge quel compito. quindi che questo Parlamento tutto rispondesse a quell'appello di don Claudio Burgio per un esercito di educatori. Sarebbe un servizio che noi potremmo fare finalmente per tutti i nostri giovani in difficoltà, altrimenti passa solo il messaggio che serve punire;

anch'io desidero approfittare dell'occasione offerta da questi emendamenti, che sosterremo tutti col nostro voto, e della presenza in Aula del ministro Nordio, per unirmi all'appello e al coro degli altri colleghi e colleghe che abbiamo già sentito.

La nostra Costituzione e il nostro ordinamento prevedono per chi sbaglia magari la perdita della libertà, ma mai la perdita della dignità. Quello che succede nelle nostre carceri è che le condizioni di vita sono tali da poter essere qualificate, secondo me, come trattamenti inumani e degradanti. Non è un caso che l'Italia sia stata condannata con la sentenza Torreggiani, ormai una decina di anni fa, e andiamo dritti in quella direzione. Tutte le colleghe e tutti i colleghi che abbiano utilizzato la prerogativa di effettuare visite nelle nostre strutture detentive sanno che quei luoghi non possono garantire alcuna forma di rieducazione e di reinserimento nella società: anzi, anzi, le statistiche ci dicono che il carcere è un luogo criminogeno. Abbiamo avuto già occasione di parlarci quando ella è venuta a rendere la sua informativa a questa Camera circa l'orientamento di una parte della maggioranza che, se oggi va ad abrogare con il voto del Senato il reato di abuso d'ufficio, ha poi introdotto almeno quindici figure di nuovi reati

purtroppo, fino ad oggi, da parte di questo Governo, un uso del diritto penale che ha aumentato i numeri, anziché diminuirli. Come diceva la collega Malpezzi poc'anzi, anche con il decreto Caivano, le statistiche ci dicono che negli ultimi tre mesi dell'anno scorso il numero dei ragazzi detenuti nelle carceri minorili è aumentato del 16 per cento. I numeri assoluti fortunatamente non sono enormi, ma comunque statisticamente c'è stato un aumento del 16 da ottobre a dicembre 2023. Delle due l'una: o decidiamo che, in linea con le sue dichiarazioni di oggi e precedenti della sua carriera di pensatore e di giurista, cominciamo seriamente a a convincerci che non c'è soltanto il carcere tra le pene, ma che ci sono tanti altri strumenti efficaci dal punto di vista della retribuzione, ma enormemente più efficaci contro la recidiva (anche lì ci vengono in soccorso i numeri), e decidiamo di adottare politiche deflattive dei numeri;

Non c'è altra possibilità: se si vuole utilizzare più carcere, le carceri devono essere fatte come si deve. Non credo che questa sia la soluzione, perché né risistemare caserme, né costruire nuove carceri sono soluzioni

è investire nella Polizia penitenziaria e soprattutto nelle figure professionali che, come ha detto molto bene la collega Malpezzi, sono davvero decisive dal punto di vista dell'impatto, per esempio gli psicologi. davanti a quest'Assemblea e con una certa convinzione: a Milano due psicologhe del carcere locale sono attualmente sotto indagine da parte della procura della Repubblica per aver fatto il loro mestiere e addirittura l'avvocata che difende l'imputata è sotto accusa. Credo che questa sia una enormità, ma certamente se già le persone le persone sono poche, non vengono pagate e poi quando fanno il loro lavoro c'è anche un pubblico ministero che le mette sotto indagine, mi pare che arriviamo a un livello completamente incontrollabile. So che lei non c'entra, ma me lo faccia dire in quest'Aula, perché

con nuove risorse su tutti gli aspetti che riguardano il tema della esecuzione della pena. Credo che tutti quanti, senza distinzione di ruolo, di partito e di Gruppo, siamo e non possiamo che essere fortemente preoccupati per la condizione in cui versano in questo momento le nostre carceri e i nostri penitenziari. Il sovraffollamento sta aumentando progressivamente e rischia di porci in rotta di collisione con l'Europa, rischiando di esporci nuovamente, come fu in passato, a sentenze della Corte europea per i diritti dell'uomo, che ci condannò, con la famosa sentenza Torreggiani,

questa situazione necessiti di un cambio di direzione di marcia significativo e visibile, perché l'inerzia, che a noi sembra in questo momento stia caratterizzando l'azione del Governo su questi punti, punti, fatalmente ci porterà verso la direzione che citavo prima, con il rischio addirittura di una nuova condanna della Corte europea per i diritti dell'uomo. L'emendamento 5.0.104 affronta uno degli aspetti sui quali noi auspichiamo - perché ovviamente facciamo il tifo - che il Governo voglia accogliere le nostre indicazioni e le nostre valutazioni. riguarda il tema degli uffici dell'esecuzione penale esterna. È già stato detto prima da qualcuno, ma tutti i giuristi lo sanno, tutti noi lo sappiamo perfettamente e lo sa meglio di me anche il Ministro: le misure alternative alla detenzione sono sanzioni, sono forme di limitazione della libertà personale, quindi sono sanzioni penali. penali. Molto spesso si pensa che l'unica sanzione penale sia la detenzione. Non è vero. Le misure alternative alla detenzione sono forme di limitazione della libertà personale, che costituiscono sanzioni a tutti gli effetti. Quelle misure, però, hanno una caratteristica, che è certificata dai dati: all'esito di quelle misure, le persone che sono state sottoposte a quelle sanzioni commettono ulteriori reati in misura molto minore di quanto non accada quando la sanzione che hanno avuto è quella della detenzione. È la famosa recidiva. E la sicurezza, tanto sbandierata e tanto cara alla destra, si tutela molto di più in questo modo che non con lo *slogan* «Buttiamoli in carcere, facciamoli marcire in galera, buttiamo la chiave». Quello è il modo, invece, per alimentare l'insicurezza, perché le persone che usciranno dal carcere, purtroppo, per le condizioni in cui versano i nostri penitenziari, ma penso anche per la natura che hanno i penitenziari, torneranno molto di più a delinquere. Quindi,

questa è un'occasione per ribadire l'invito ad andare con convinzione in quella direzione, se vogliamo risolvere il problema delle nostre carceri e se vogliamo affrontare in maniera seria il problema della sicurezza nel nostro Paese.

Prima però di intervenire nel merito, mi sia consentito di ringraziare un nostro collega che per ragioni di salute non può essere con noi. Questa battaglia che il Partito Democratico e il Senato stanno affrontando sul tema carceri è coerente con un impegno costante che nella passata legislatura, ma anche in questa, nonostante l'impedimento che non gli permette di stare con noi, il nostro collega Franco Mirabelli ha condotto e conduce su questi temi.

grande sincerità, ma soprattutto con grande senso della realtà ha definito non solo drammatica - lo vediamo - la situazione delle carceri italiane, ma soprattutto ha detto una cosa che non ha una soluzione alle viste. Ministro, eravamo insieme qualche giorno fa, sia pure per un'occasione particolare, al carcere Regina Coeli e ho ascoltato le sue prese di posizione che rivelano un'attenzione e anche forse, se posso intuire, un'angoscia personale rispetto alla situazione del carcere, al fatto che le proiezioni

al di là delle angosce e delle preoccupazioni, questa realtà richiede un intervento immediato. Come intendete, qui ed ora, Ministro, Governo, dare delle risposte immediate al fatto che i detenuti oggi nelle carceri italiane sono 60.000

delle iniziative per rendere meno pesante il sovraffollamento". Al contrario, voi avete introdotto reati che porteranno ad aumentare il numero dei detenuti, anche per reati minori, i quali non dovrebbero magari stare in carcere. Invece di intervenire con misure di lotta al sovraffollamento, fate l'esatto contrario. E non è un problema - come ho sentito dire - costruire nuove carceri, che sono di là da venire; è un problema del qui e ora. State anche smantellando il tema della giustizia riparativa, anche culturalmente lo state facendo. Siete intervenuti per colpire qualsiasi possibilità di pena alternativa. Invece il Partito Democratico - e finisco, ma ho voluto dire adesso generalmente queste cose - vi chiede di intervenire subito. Questo emendamento prevede un intervento particolare per portare a 500 le unità che possono intervenire dal punto di vista psicologico. Guardi, è la stessa cosa che ha detto ieri il DAP. Mi permetta, Ministro, è la stessa cosa che ha detto a questo Parlamento l'altro giorno Sergio Mattarella ed è la stessa cosa che chiedono tante persone. È umanità ed è rispetto della Costituzione.

Signora Presidente, restando chiaramente in tema di investimenti e ponendo una particolare attenzione alle donne detenute e chiaramente ai figli minori, chiediamo un'implementazione del numero degli istituti di custodia attenuata per le detenute madri. Purtroppo in Italia ve ne sono soltanto cinque e quasi tutti nel Nord Italia. Infatti ce n'è uno a Milano, uno a Torino e uno a Venezia; ne abbiamo uno in provincia di Cagliari e un altro in provincia di Avellino. Il Sud ne risulta assolutamente scoperto. Quindi invitiamo a votare a favore di questo emendamento. Medesimo e identico discorso

Signora Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole e per richiamare l'attenzione del Ministro e dell'Assemblea sul fenomeno dei bambini che crescono nelle carceri; questa è veramente un'altra questione che proprio non si può accettare, signor Ministro. Basta parlare con la Polizia penitenziaria, basta fare due chiacchiere con loro. Mi è successo alla "Dozza" a Bologna, dove peraltro c'è un angolo del carcere che è stato colorato, per quanto si possa rendere accettabile uno spazio di quel genere. Mi diceva una genere. Mi diceva una donna della Polizia penitenziaria che, quando si aprono i cancelli, i bambini tendono a correre verso il cancello che si apre, ma ovviamente devono essere rimessi dentro. Io penso che un Paese come il nostro, un Paese civile,

Signora Presidente, signor Ministro torniamo ancora una volta sulla questione dei bambini in carcere. Noi lo vogliamo dire con grande chiarezza in quest'Aula. I bambini non devono stare in carcere. Mai più bambini in carcere. Vorremmo che, oltre alla lacrima visibile, di circostanza, quando si scopre che c'è un bambino in carcere, come recentemente accaduto nella mia città,

a lei, signor Ministro, anche per il tramite della Presidente. Signor Ministro, ella più volte su questo argomento si è commosso, si è indignato, proponendo una serie di impieghi suppletivi, alternativi, per incrementare l'edilizia carceraria. Ora, a parte il fatto che che ci vorranno anni per realizzare questo tipo di interventi, la questione vera è che la maggioranza alla quale lei appartiene si disinteressa e non ritiene di doversi interessare a che cosa succede nelle carceri: cioè al trattamento dei detenuti, con tutte le funzioni che ne discendono. Questo emendamento, in particolare, propone di incrementare il fondo destinato alle case famiglia, che ha proprio a che vedere con la questione dei bambini che non devono stare in carcere. Noi proponiamo che questo fondo sia incrementato di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Ancora una volta, si tratta di scegliere dove mettere i soldi e a cosa dare la priorità. Non comprendiamo davvero come non si possa accogliere questo emendamento.

questo è un emendamento che stanzia 20 milioni di euro per la ricerca e 20 milioni aggiuntivi per la manutenzione delle strutture in cui i minori si trovano e per le residenze. Lo dico perché il luogo dove ci si trova è molto importante. Ci siamo occupati negli emendamenti precedenti della dotazione dell'organico, che come sappiamo è una delle questioni più spinose della situazione carceraria, sia

se si ha l'idea che i giovani e i ragazzi debbano essere recuperati. È una nostra missione: sono centinaia di migliaia i ragazzi in situazioni di fragilità nel nostro Paese. Approfitto della discussione di questo emendamento, Presidente, avendo l'opportunità di parlare

Si fanno tante classifiche per misurare il grado di civiltà e di democrazia di un Paese, ma c'è un dato che dà la cifra ed è come vengono considerati i più fragili e i più vulnerabili. Gli ultimi degli ultimi sono i membri della popolazione carceraria: è lì che spesso si fa la differenza anche su quella che è la prospettiva che noi ci diamo. Il dato sul malessere e sulla salute dei detenuti nelle carceri nel nostro Paese è assai preoccupante e questo ci dovrebbe spingere, da una parte, ad aumentare il personale sanitario,

in un carcere. Non può stare nemmeno un paziente psichiatrico in un carcere *(Applausi)*, non è quello il suo posto. Sappiamo che i problemi vengono da lontano, ma abbiamo il dovere di affrontarli, anche con una certa urgenza, visto che purtroppo i numeri ci riportano ad una realtà che non è più allontanabile dal nostro pensiero e dalle nostre azioni.

Signor Presidente, vorrei porre l'attenzione su un tema che sappiamo stare a cuore al Governo, che è il tema delle strutture penitenziarie per i minorenni. già stato detto prima, voi avete approvato il decreto-legge Caivano, che ha profondamente innovato la giustizia penale minorile, purtroppo, dal nostro punto di vista, mettendone in discussione i capisaldi e avvicinandola pericolosamente ai principi che governano, invece, la giustizia penale per adulti, in questo modo scardinando gli obiettivi, le finalità, i principi e l'ispirazione che devono muovere la giustizia penale minorile, che non può essere solo quella della punizione, ma deve essere anzitutto quella del recupero dei ragazzi. Tutto questo noi lo avevamo denunciato come rischio e ce l'avevano detto anche gli auditi in quella circostanza, che avrebbe portato a un aumento dei detenuti minori nelle carceri per minorenni, in una condizione

di saturazione dei nostri penitenziari minorili e, per effetto di quelle norme, ci sarebbe stato un incremento. Questo purtroppo è avvenuto e i dati recenti pubblicati da «Il Sole 24 Ore» dicono che, ad oggi, per effetto delle norme del decreto-legge Caivano, sono aumentati del 16 per cento i detenuti nei penitenziari minorili. Questo sta provocando, inevitabilmente, un problema anche nei nostri penitenziari minorili. Credo che questo sia un tema che deve essere affrontato poiché ineludibile e riguarda quantomeno e anzitutto la ristrutturazione, la messa a norma e la sistemazione dei padiglioni e degli spazi per le strutture penitenziarie per i minorenni. So che il sottosegretario Ostellari, che ha seguito questa materia, è sensibile alla questione, mi dispiace che non si dia un segnale, quantomeno in questa circostanza, su un argomento su un argomento che penso meriterebbe invece maggiore attenzione. Non pretendiamo che venga accolto *in toto* un emendamento che invita a spendere soldi che evidentemente in questo momento non ci sono.

all'intera maggioranza. Come prima è stato fatto con un emendamento della collega Rossomando, mi dichiaro disponibile, se c'è questa disponibilità da parte della maggioranza e del Governo, a trasformare anche questo nostro emendamento in ordine del giorno, perché è un modo per essere concordi sulla necessità di intervenire in proposito.

Vorrei dire che questo nostro emendamento pone il problema del finanziamento dell'architettura penitenziaria.

di trattamento, a un'idea di applicazione dell'articolo 27 della Costituzione, a una concezione della pena (quando è detentiva in carcere) come recupero, come rieducazione, come reinserimento. Oggi nelle carceri, sia quelle fatiscenti (e sono tante), sia quelle di più recente costruzione, questi principi non vengono minimamente tenuti in considerazione. Allora, secondo noi, mentre si deve combattere contro il sovraffollamento con provvedimenti deflattivi davvero efficaci, al tempo stesso per chi sconta la pena dentro le carceri occorre prevedere

che hanno da scontare soltanto ancora pochi mesi, magari di lavorare all'esterno e non di farli tornare a dormire in carcere, come avete fatto bocciando le nostre richieste di deroga per far tornare il regime dei semiliberi che, durante il Covid, uscivano e non tornavano a dormire. *(Applausi)*. Bisogna fare in modo che le carceri siano umane e l'architettura carceraria è un pezzo di questa concezione. Noi non siamo tra quelli che dicono: buttiamo via la chiave, marciscano in galera. Noi pensiamo davvero che la pena, quando è giusta e quando deve esserci, debba essere rieducativa, anche perché un detenuto che esce rieducato poi non torna a delinquere, come dicono le statistiche sulle recidive. Pertanto, è necessario investire in umanità è investire in sicurezza.

Per esempio, si sta riducendo il numero delle telefonate ai propri familiari, adesso si stanno riducendo le ore di apertura delle sezioni, perché c'è un problema di personale. La vigilanza dinamica è un problema problema serio perché manca personale di Polizia penitenziaria, tuttavia si costringeranno i detenuti a stare ancora di più chiusi in celle sovraffollate per tante ore al giorno. Questo aumenterà la tensione nelle carceri, non la diminuirà, proprio mentre c'è stata una sentenza della Corte costituzionale che richiama tutti noi. Se il Parlamento non lo facesse, la Corte dice che lo faccia il DAP richiama tutti noi a garantire anche l'affettività dentro le carceri. Signor Presidente, intervenire sull'architettura significa intervenire su una concezione della pena e del trattamento penitenziario coerente con princìpi costituzionali.

se almeno una volta, durante il loro mandato, iniziato prima o dopo, si sono presi un po' di tempo per fare una visita in una delle carceri presenti su tutto il territorio nazionale. A me è capitato la settimana scorsa, ma ero già stata circa un anno fa a Torino, nella sezione femminile, che mi aveva impressionata particolarmente per gli spazi angusti poi mi avevano anche riferito che tutto sommato, rispetto ad altre sezioni, non erano neanche così angusti. Mi domando se noi, che viviamo nelle nostre case spaziose, con camere, salotti, cucine, terrazzi, balconi, abbiamo mai provato ad immedesimarci nella vita di persone che devono passare giorni, settimane, mesi, anni dopo anni all'interno di spazi angusti, con finestre piccolissime, a volte anche in sezioni o padiglioni che solo per qualche giorno all'anno vengono illuminati direttamente

alla base di un pendio montuoso, in una zona che riceve il sole solo in una direzione per alcuni giorni nei mesi invernali

vorrei che cercassimo tutti di capire che cosa vuol dire vivere lì dentro per anni, in spazi angusti e dovendo dividere ogni spazio vitale costantemente con qualcun altro, senza avere mai un

scontando una pena, ma c'è anche chi si ritrova lì in attesa di giudizio e quindi, per la nostra legislazione, con presunzione di innocenza. Chiederei che tutti insieme facciamo una riflessione troviamo una soluzione e le risorse adeguate perché ci siano misure detentive alternative, quando questo è consentito, ma comunque quando invece siamo obbligati alla detenzione, di fare in modo che ci siano spazi umani, ci siano docce che non abbiano la muffa alle pareti, docce che abbiano sempre l'acqua calda, celle che abbiano soluzioni individuali per chi lo preferisce o comunque spazi adeguati per una corretta esistenza e per la tutela dei diritti umani. Credo che questo sia il minimo che un Paese che si voglia ritenere civile debba consentire ai propri cittadini.

che non ci possa essere un atteggiamento di rassegnazione rispetto allo stato di emergenza in cui versano le carceri italiane. È chiaro che non è una responsabilità di questo Governo in particolare: è un'emergenza che ci portiamo appresso da decenni, rispetto alla quale, però, abbiamo una responsabilità, se vogliamo veramente rispettare la Costituzione, che richiede la finalità rieducativa della pena. Le carceri oggi sono in condizioni disumane. C'è un problema di sovraffollamento, che non si risolve solo attraverso la misura della riduzione della custodia cautelare. Servono nuovi edifici, serve togliere la paura della firma. Al Ministro mi sento di chiedere di valutare con attenzione il contenuto di questo emendamento, perché mi sembra di grande buon buon senso, è uno scatto in avanti, senza addossare la responsabilità agli uni o agli altri, ma facendo un gioco di squadra, per dare qualche segnale a coloro che si trovano dentro le carceri italiane, anche a coloro che ci lavorano. Il sovraffollamento, infatti, è un problema per i detenuti, ma lo è anche per la Polizia penitenziaria. *(Applausi)*. Io credo allora, signor Ministro, che questo emendamento sia di grande buon senso e che lei abbia l'esperienza, l'umanità e la

a una ricorrenza che una legge dello Stato ha fissato per il 10 febbraio di ogni anno. È la legge che ha istituito il Giorno del ricordo nel 2004, per onorare la memoria di coloro che hanno perso la vita nell'orrore delle foibe e di quanti hanno dovuto affrontare il dolore e le sofferenze dell'esodo giuliano dalmata,

il dramma delle foibe, il dramma soprattutto di chi era rientrato in Italia sperando di essere abbracciato come figlio esule della propria Nazione, della propria Patria,

pur avendola sempre saputa. Faccio parte di una minoranza che la conosceva perché tramandata dagli amici, dai genitori

legami ideologici con i comunisti di Tito che avevano perpetrato quegli orrori, ma fu una responsabilità molto più ampia.

quella drammatica realtà con il rispetto che merita e con la parola "ricordo", che non a caso fa parte del

L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla vicenda di Ilaria Salis, detenuta in Ungheria».

Signor Presidente, onorevoli senatori, mi scuso per il ritardo, ma ho partecipato all'ennesimo identico dibattito nell'Aula di Montecitorio. Sto seguendo, insieme al Ministero internazionale e a tutti i nostri diplomatici, 2.405 casi di cittadini italiani detenuti all'estero.

Ho detto alla Camera che l'Italia è la Patria di Cesare Beccaria. L'Italia è la culla del diritto l'azione del Governo è sempre e comunque ispirata alla difesa e al rispetto del diritto italiano, del diritto comunitario e del diritto internazionale. Il garantismo ispira il nostro agire per tutti i detenuti italiani all'estero (ripeto: 2.405), che seguiamo costantemente per tutelare i loro diritti. Indipendentemente dall'essere detenuto in attesa di giudizio (pregiudicato o incensurato), condannato in primo grado, condannato in via definitiva, c'è soltanto una regola che deve essere rispettata, quella della tutela della dignità della persona. ci siamo sempre battuti e continueremo a batterci. Lo dico anche perché ho l'onore di guidare una forza politica che del garantismo ha fatto una sua bandiera. Quindi, sono assolutamente convinto della necessità di impegnarci sempre e comunque per tutelare i diritti di ogni persona. Fin dai primi giorni della sua detenzione, ben prima che diventasse oggetto di polemiche politiche, i nostri diplomatici si sono impegnati per far sì che venisse sempre e comunque rispettato il caso della signora Ilaria Salis. Vi devo illustrare i fatti, perché poi possiate giudicare, nella vostra coscienza e politicamente, se c'è stato o meno interesse, interesse, da parte della diplomazia italiana, nei confronti di questa detenuta. Non posso raccontarvi di tutti gli altri 2.404 detenuti, perché ci vorrebbe parecchio tempo. Il 13 febbraio 2023 la procura di Budapest ha informato l'ambasciata d'Italia che la signora Ilaria Salis era stata posta in stato di fermo due giorni prima, con l'accusa di violenza armata di gruppo. L'aggressione di cui la signora Salis è accusata sarebbe avvenuta al termine di una manifestazione politica di estrema destra. La connazionale, sempre secondo l'accusa, apparterrebbe a gruppi organizzati che avrebbero pianificato l'aggressione di alcuni militanti presenti alla manifestazione. Un'indagine è in corso anche in Germania su soggetti di nazionalità tedesca, alcuni dei quali destinatari di mandati di cattura nazionali per reati commessi nella stessa circostanza. La signora Salis è stata rinviata a giudizio ed è attualmente detenuta in carcere a Budapest; la richiesta da parte della procura è di una pena detentiva di undici anni. L'ambasciata d'Italia si è attivata immediatamente per fornire ogni possibile assistenza alla signora Salis e ai suoi familiari, con cui ha intrattenuto un intenso dialogo. Ha effettuato frequenti visite consolari in carcere ed è intervenuta per venire incontro alle richieste della connazionale rispetto alle sue condizioni detentive. Il 14 febbraio si è svolta la prima udienza davanti al giudice per le indagini preliminari, cui ha assistito anche un funzionario dell'ambasciata, che ha incontrato la signora Salis e il suo legale. Durante l'udienza è stata accolta la richiesta dell'accusa di custodia cautelare in carcere. La signora Salis è stata invece prosciolta da una seconda imputazione per un'altra aggressione, poiché era stato comprovato che, al momento dello svolgimento dei fatti di quella aggressione, non si trovava in Ungheria. L'autorità giudiziaria ungherese ha poi, con successivi provvedimenti, prorogato la custodia cautelare della signora Salis, misura consentita dalla legge ungherese per indagini relative a reati di violenza di gruppo. Il giorno dopo la prima udienza, il 15 febbraio 2023, l'ambasciata ha riferito al signor Roberto Salis del colloquio con la figlia. Gli ha assicurato ogni collaborazione per inviarle beni e denaro e lo ha informato dell'assistenza consolare che le nostre sedi possono fornire ai detenuti italiani all'estero. Il 19 febbraio la signora Salis ha scritto all'ambasciata per descrivere le sue condizioni detentive, lamentando in particolare cimici nel letto. L'ambasciata ha contattato subito il legale della connazionale per una richiesta di cambio di cella; richiesta accolta. Il 3 marzo la signora Salis ha confermato all'ambasciata di essere stata trasferita in una cella senza cimici, ma ha riferito altri problemi: la visita del medico non ancora ottenuta, la mancanza dell'ora d'aria e di strumenti per la pulizia della cella. L'ambasciata ha segnalato tempestivamente al penitenziario le varie problematiche, chiedendone la risoluzione. Con provvedimento del 9 marzo 2023, la procura generale di Budapest ha inizialmente imposto alla connazionale un regime di detenzione fortemente restrittivo. Il provvedimento della procura proibiva i contatti della signora Salis con i genitori e non consentiva nemmeno quelli con due cittadini italiani, indicati dalla signora Salis come persone di riferimento nella richiesta inoltrata tramite il proprio legale ungherese. L'ordinanza non consentiva neppure i contatti richiesti con l'avvocato italiano. Le possibilità di comunicazione con l'esterno, perciò, erano in un primo momento limitate al solo legale ungherese della signora Salis e all'ambasciata d'Italia a Budapest. Tale condizione è stata confermata anche da una lettera del 15 marzo 2023, con la quale la signora Salis informava del divieto di contattare i genitori e i legali italiani e chiedeva all'ambasciata di farlo, cosa che è avvenuta nella stessa giornata. Sabato 16 marzo l'ambasciata è riuscita ad ottenere, per il successivo mercoledì, l'autorizzazione a effettuare la prima visita consolare in carcere, chiesta già a febbraio. La visita è stata appunto effettuata il 20 marzo. In tale occasione, il personale dell'ambasciata ha consegnato alla signora Salis indumenti e altri generi di prima necessità e ha raccolto le istanze della connazionale in merito alle condizioni di detenzione e ai suoi contatti con l'esterno. La signora Salis ha lamentato il fatto che le fossero impediti i contatti con i genitori, l'avvocato in Italia e le persone da lei indicate come punti di riferimento, nonché il fatto di trovarsi da sola in cella. La signora Salis ha comunque confermato di disporre dei fondi necessari per il proprio sostentamento e di poter comunicare regolarmente con il proprio avvocato ungherese. Ha inoltre manifestato l'intenzione di chiedere il trasferimento in Italia ed espresso il desiderio di sfruttare il tempo della detenzione per prepararsi a un concorso pubblico. L'ambasciata ha subito inviato alla madre la richiesta di libri. Grazie all'azione di sensibilizzazione condotta dalla nostra sede nei confronti delle autorità ungheresi, la signora Salis ha ottenuto un miglioramento delle condizioni detentive: dalla concessione dell'ora d'aria alle condizioni igieniche e all'effettiva ricezione del denaro inviatole, come lei stessa ha confermato in una lettera del 24 marzo. Anche durante la seconda visita consolare in carcere, svoltasi il 5 aprile, il personale dell'ambasciata ha consegnato alla signora Salis un pacco con indumenti e generi di prima necessità e ha nuovamente parlato con lei del suo stato di salute e delle condizioni detentive. In una lettera del 19 aprile, la signora Salis ha informato l'ambasciata di essere stata spostata, il giorno 13 aprile, in una cella più spaziosa e condivisa con altre due detenute. Poiché la connazionale lamentava scarse condizioni igienico sanitarie, l'ambasciata ha contattato il penitenziario ottenendo di spostare nuovamente la signora Salis in un'altra cella. Il 26 aprile il vice capo missione, responsabile dell'ufficio consolare, ha avuto una videoconferenza con i genitori della signora Salis, i legali ungheresi italiani e le persone indicate dalla detenuta come punti di contatto. Il 9 maggio la detenuta ha chiesto all'ambasciata aiuto nel disbrigo di pratiche relative al concorso cui intende partecipare. L'ambasciata ha inoltrato la richiesta al contatto indicato dalla signora Salis. Il 18 maggio si è svolta la terza visita consolare in carcere. In tale occasione, è stato possibile consegnare alla detenuta un pacco contenente libri e altro materiale didattico per la preparazione al concorso. In questa occasione, la signora Salis ha confermato che le problematiche precedentemente sollevate erano state risolte. Ha riferito della sua partecipazione ad attività formative organizzate dalla struttura, mentre ha comunicato che il ricorso per poter avere contatti con i genitori era stato respinto. Il 9 giugno il vice capo missione ha assistito a un interrogatorio della detenuta. Il 13 giugno 2023 lo stesso funzionario ha ricevuto in ambasciata il signor Roberto Salis, il compagno e due conoscenti della signora Salis. In tale occasione ha ribadito la piena disponibilità della rappresentanza ad attivarsi in qualsiasi momento per assistere la connazionale. Il giorno 5 luglio il personale dell'ambasciata ha effettuato una quarta visita in carcere e ha consegnato un nuovo pacco con indumenti e libri richiesti. La detenuta ha lamentato il fatto che da quasi un mese non riceveva il consueto bonifico, con la conseguenza impossibilità di acquistare beni di prima necessità. Terminata la visita, l'ambasciata si è attivata per risolvere il problema. Il 21 luglio ho inviato una nota verbale alla procura generale, chiedendo un incontro con la procura generale per discutere del regime di detenzione della signora Salis. Il 26 luglio il vice capo missione e l'addetto consolare hanno incontrato alti funzionari della procura generale, la direttrice generale per la supervisione delle indagini, il capo del dipartimento affari internazionali e del dipartimento monitoraggio della legislazione sull'applicazione delle leggi penitenziarie. L'intervento era stato concordato con il signor Roberto Salis e con i legali in vista della successiva udienza. Nel rimarcare la grande attenzione per il caso Salis, l'ambasciata è tornata a sensibilizzare le controparti ungheresi sulle condizioni detentive della signora. In particolare, sono state evidenziate l'impossibilità per la nostra connazionale di comunicare con l'esterno e le esigenze alimentari della detenuta. A questo intervento, l'ambasciata ha fatto seguire, il 3 agosto, un'apposita comunicazione all'istituto penitenziario per ribadire la necessità di attuare la dieta prescritta dal medico alla signora Salis. L'11 agosto si è svolta una nuova udienza davanti al giudice per le indagini preliminari, che ha ulteriormente esteso il fermo cautelare. Analogamente a quanto fatto in precedenza, l'addetto consolare dell'ambasciata ha partecipato all'udienza e ha incontrato la signora Salis e il suo legale. In una missiva del 29 agosto all'ambasciata, la signora Salis si è lamentata della mancanza d'aria nella cella a causa della scarsa apertura della finestra e dell'afa. A seguito della lettera, l'ambasciata ha contattato il penitenziario per richiedere un nuovo cambio di cella. La signora Salis ha informato l'ambasciata che la dieta veniva rispettata regolarmente e in una lettera del 1° settembre ha riferito che il regime di detenzione era stato significativamente allentato. Alla connazionale venivano in particolare consentiti contatti regolari con i genitori attraverso visite e chiamate via Skype, passi avanti ottenuti proprio grazie alla costante sensibilizzazione della nostra ambasciata. Il 12 ottobre i genitori della signora Salis sono stati nuovamente ricevuti in ambasciata insieme agli avvocati italiani, al compagno e un'amica della connazionale. La quinta visita consolare si è svolta il giorno 25 ottobre. Oltre alla consegna del pacco inviato dai genitori e dagli amici, i funzionari dell'ambasciata hanno avuto un nuovo colloquio con la signora Salis. Subito dopo la visita, il vice capo missione e l'addetto consolare hanno incontrato il nuovo direttore degli istituti penitenziari di Budapest per ribadire la massima attenzione al caso e l'importanza di garantire condizioni carcerarie dignitose e rispettose dei diritti della detenuta. In particolare, hanno sollecitato - come richiesto dalla stessa signora Salis - che fosse effettuato un cambio di lenzuola regolare e che il regime dietetico venisse confermato ed esteso. L'udienza del 14 novembre ha confermato la proroga della custodia cautelare in carcere. Il 21 novembre i genitori della signora Salis sono stati ricevuti in ambasciata per un nuovo incontro sugli aggiornamenti processuali e difensivi. In quell'occasione hanno confermato la possibilità di contatti regolari con la figlia attraverso visite e chiamate via Skype. Il 13 dicembre l'ambasciata ha effettuato la sesta visita consolare presso il penitenziario. In questa occasione la signora Salis ha sottolineato la necessità di visionare gli atti del processo opportunamente tradotti e i video a suo carico. Il 19 dicembre l'ambasciata ha sollecitato entrambe le questioni con una nota verbale al Ministero degli esteri ungherese. Il riscontro ricevuto il 12 gennaio di quest'anno ha indicato le modalità di accesso ai fascicoli relativi a procedimenti penali e, in vista della prima udienza processuale e considerando quindi la chiusura delle indagini, il 22 gennaio 2024, in occasione del Consiglio affari esteri dell'Unione europea, ho sollevato il caso con il Ministro degli esteri ungherese in occasione di un incontro bilaterale che ho appositamente chiesto. Al Ministro ho sottolineato che la signora Salis lamentava di avere difficoltà nell'accesso agli atti processuali tradotti e ai video prodotti come prova a suo carico. Ho ricordato che la detenuta era stata lungamente sottoposta a un regime di custodia cautelare che ne aveva limitato fortemente le possibilità di interazione con l'esterno e ho sottolineato che il Governo italiano esige il rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalle norme europee, in sintonia con la nostra civiltà giuridica. Ho inoltre sottolineato l'auspicio di una revisione del regime di custodia cautelare concedendo alla detenuta misure alternative. A questo fine ho consegnato al mio collega ungherese un documento scritto che conteneva tutte le cose che vi ho appena riferito. Ancora non era esplosa la polemica politica e il 23 gennaio il ministro Nordio ha ricevuto il signor Roberto Salis. Nel corso del colloquio, il Ministro della giustizia ha suggerito l'opportunità di avanzare domanda di arresti domiciliari in Ungheria. Si tratta - a nostro giudizio - di una questione giuridica dirimente, perché la concessione di misure cautelari alternative alla detenzione, che deve essere richiesta dai legali e disposta dall'autorità giudiziaria ungherese, è condizione necessaria per invocare l'attivazione della decisione quadro n. 829 del 2009, che consente il reciproco riconoscimento tra i Paesi membri dell'Unione europea delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione. In tre circostanze l'avvocato della signora Saris aveva presentato istanza di misure alternative al carcere, ma in tutti e tre i casi era stato chiesto che la misura venisse applicata direttamente in Italia. Le istanze sono state respinte dal magistrato ungherese. Il ministro Nordio ha invece sottolineato al signor Salis come un'istanza di misura alternativa in Ungheria abbia maggiori possibilità di essere accolta dall'autorità giudiziaria ungherese. Soltanto dopo la concessione di una misura alternativa in Ungheria, sarà possibile proporre un'ulteriore istanza per ottenere l'applicazione di tale misura in Italia, ai sensi della suddetta decisione quadro europea. Tutto ciò, onorevoli senatori, per dire che si possono fare tante dichiarazioni, ma poi bisogna agire utilizzando gli strumenti giuridici che sono a disposizione. Per questo ho detto che noi rispettiamo il diritto italiano, europeo e internazionale. Il 24 gennaio l'ambasciatore ha effettuato una visita consolare in carcere alla signora Salis, ha ribadito ancora una volta la massima attenzione con la quale l'ambasciata segue il caso e reitirato la disponibilità a sostenere future richieste inoltrate della difesa in merito alla richiesta di misure alternative al carcere. Nell'udienza del 29 gennaio 2024, la signora Salis ha respinto le accuse dichiarandosi innocente. L'avvocato della signora Salis ha rilevato durante l'udienza la mancanza della traduzione degli atti di accusa in italiano e la mancata visione del video di sorveglianza, lamentando dunque una non piena informazione e comprensione, da parte della signora Salis, del capo di imputazione. Il suo legale non ha presentato domanda di misure cautelari alternative al carcere in Ungheria, contrariamente a quanto era stato suggerito dal ministro Nordio. La prossima udienza è stata calendarizzata per il 24 maggio e in tale occasione sarà chiamata a testimoniare anche la parte lesa. Nei colloqui che abbiamo avuto, abbiamo sollecitato la politica a far sì che venissero inviati messaggi Le immagini della prima udienza processuale, quella del 29 gennaio, con l'imputata condotta in aula in catene hanno giustamente colpito tutti noi. In una lettera al suo avvocato italiano, ricevuta pochi giorni prima dall'ambasciata, la signora Salis aveva fatto una serie di considerazioni sulla situazione processuale e sulle condizioni carcerarie, e tra le numerose questioni aveva menzionato anche l'uso delle catene in udienza. Ma, dal momento che è pratica purtroppo comune e prevista dalla normativa locale nel caso dei reati più gravi connessi a violenza, lo stesso avvocato ungherese della detenuta non aveva mai incentrato su questo specifico aspetto una richiesta di intervento da parte della ambasciata. L'esibizione delle catene in aula dell'imputato con le immagini trasmesse in televisione ha avuto un forte impatto. Quindi, nonostante la mancata richiesta da parte dell'avvocato ungherese, il Governo è intervenuto, e questo perché la traduzione in carcere con catene ai polsi e ai piedi non è in linea con lo spirito delle norme europee. La direttiva n. 343 del 2016 prevede, infatti, che gli Stati membri adottino misure appropriate per garantire che gli indagati e gli imputati non siano presentati come colpevoli in tribunale o in pubblico attraverso il ricorso a misure di coercizione fisiche, pur prevedendo che si possano adottare misure coercitive necessarie per ragioni di sicurezza legate al caso di specie. Proprio per questo motivo ho immediatamente chiesto con una dichiarazione pubblica al Governo ungherese di vigilare e intervenire affinché venissero rispettati i diritti della cittadina italiana

e al nostro ambasciatore di fare un passo ufficiale presso le autorità di Budapest. Il 30 gennaio il segretario generale della Farnesina ha quindi incontrato l'incaricato d'affari dell'ambasciata ungherese - l'ambasciatore non era a Roma, quindi lui era il più alto in grado - per ribadire la grande attenzione con cui il Governo italiano segue la vicenda. L'ambasciatore Guariglia ha espresso la protesta del Governo italiano per le condizioni in cui la signora Ilaria Salis è stata detenuta e viene trattenuta durante le udienze

Il segretario generale Guariglia si è inoltre soffermato sull'assoluta necessità che alla signora Salis e ai suoi legali siano garantiti l'accesso alla traduzione in italiano degli atti di accusa così come già richiesto dalla difesa - e la visione del video di sorveglianza alla base dell'imputazione, per assicurare il pieno godimento del diritto alla difesa e un equo processo. Nella stessa giornata del 30 gennaio 2024, il nostro ambasciatore a Budapest ha ricevuto i genitori, il compagno, alcuni congiunti e il legale della signora Salis. I genitori della signora Salis sono poi stati accolti dall'ambasciatore il giorno successivo. Su mia istruzione, l'ambasciatore l'ambasciatore Jacoangeli, nel pomeriggio del 30 gennaio, ha incontrato il Ministro della giustizia ungherese per reiterare le rimostranze circa le condizioni di carcerazione della connazionale e il trattamento riservato alla signora Salis in aula. Il Ministro ha comunicato di aver richiesto al procuratore generale una relazione dettagliata sulla vicenda. In seguito a questo incontro, la signora Salis ha ricevuto la visita del procuratore capo, di una psicologa e di una educatrice. La connazionale ha poi riferito, in una successiva lettera pervenuta all'ambasciata il 1° febbraio, che il verbale dell'incontro propostole per la firma era solo in ungherese; l'ambasciata ha subito comunicato all'avvocato italiano il contenuto della lettera e ha inviato alle autorità ungheresi una nota verbale con la richiesta di una copia del documento firmato dalla signora Salis. Il presidente del Consiglio Meloni ha affrontato il caso di Ilaria Salis con il primo ministro ungherese Viktor Orban in due occasioni: la prima al telefono il 30 gennaio, la seconda a margine dei lavori del Consiglio europeo il 2 febbraio. Nel rispetto dell'autonomia dei giudici, che ovviamente esiste anche in Ungheria, ha chiesto che vengano riservati alla nostra connazionale un trattamento di dignità e rispetto e un giusto processo. Ho ribadito tale auspicio al Ministro degli esteri ungherese, da me di nuovo incontrato a Bruxelles il 1° febbraio. Il 5 febbraio il ministro Nordio ed io abbiamo ricevuto in due incontri successivi il signor Roberto Salis, che ha fatto due richieste: una missiva del Governo italiano alla magistratura in ungherese per favorire la concessione di una misura cautelare alternativa alla detenzione e l'ipotesi che tale misura possa essere eseguita presso l'ambasciata. Abbiamo detto al signor Salis che, qualora i Ministeri dell'interno e della giustizia avessero autorizzato una tale ipotesi, io personalmente non mi sarei affatto opposto. opposto. Ho detto che servivano le autorizzazioni dei Ministeri dell'interno e della giustizia, atteso che l'ambasciata non è una casa privata, ma è un edificio pubblico e pertanto, dovendo esserci un detenuto che noi non conosciamo, non non possiamo lasciarlo circolare liberamente dentro l'ambasciata. Quindi, servivano dei locali appositamente predisposti e serviva un incremento dei carabinieri nell'ambasciata per i necessari controlli e la la necessaria tutela del detenuto, perché sempre di detenuto si tratta, anche se agli arresti domiciliari, dei quali l'Italia ha la responsabilità, in quanto l'ambasciata che è territorio italiano, ma anche di evasione, quindi del tutto responsabile. Anche oggi i detenuti agli arresti domiciliari hanno il controllo da parte delle Forze dell'ordine, ma si tratterebbe di una situazione molto Il ministro Nordio ha illustrato le ragioni di diritto e di fatto, per cui la richiesta di sostituzione della misura cautelare presso l'ambasciata italiana non è possibile. L'ambasciata non è luogo idoneo all'esecuzione di misure coercitive, non ha né la struttura, né la legittimazione a sostituirsi a un domicilio privato come luogo di detenzione. Non è una presa di posizione contraria per principio, veramente quasi impossibile tenere un qualsiasi detenuto all'interno di un'ambasciata; ne abbiamo 2.405 non tutte le ambasciate sono attrezzate per ospitare, eventualmente, detenuti italiani che chiedessero, quelli in attesa di giudizio o anche quelli condannati, di scontare la pena dentro l'ambasciata d'Italia e non nel carcere di altri Paesi. La situazione La situazione dei marò, citata come termine di paragone dal signor Salis, non è in realtà equiparabile, perché il reato contestato ai marò era stato commesso su nave italiana in acque internazionali. L'Italia ha da subito contestato la giurisdizione delle autorità indiane, dando vita a una controversia internazionale in cui ha poi prevalso. Era in discussione l'immunità di due militari italiani nell'esercizio delle proprie funzioni. L'Italia riteneva, cioè, che l'esercizio da parte indiana della propria giurisdizione violasse gli obblighi internazionali di rispettare l'immunità dei pubblici ufficiali di Stati stranieri un tribunale internazionale ha poi dato ragione all'Italia proprio sulla base del principio per cui gli Stati non hanno giurisdizione su altri Stati. Diverso appare il caso della signora Salis, in cui l'Italia non contesta, né può contestare la giurisdizione ungherese, perché ogni Stato ha diritto di esercitare la giurisdizione penale per reati commessi sul proprio

indiano, ma su una nave italiana, e quindi sul territorio italiano, e in acque internazionali. Diversamente, l'ipotetico reato che viene contestato alla signora Salis è stato commesso in Ungheria. Questa è la differenza: non è questione di gravità del reato, ma è questione di competenza Il ministro Nordio ha inoltre rilevato che un'interlocuzione epistolare tra il Dicastero italiano e un organo giurisdizionale straniero sarebbe irrituale e irricevibile. La decisione sullo stato di libertà dell'indagato compete solo al giudice ungherese. Se il documento richiesto fosse una semplice spiegazione, il magistrato ungherese potrebbe rispondere che già conosce la nostra legge; se invece fosse una surrettizia richiesta di convertire la custodia cautelare in carcere in arresti domiciliari, allora sarebbe una interferenza.

ottengono l'effetto contrario a quello desiderato, e cioè si fanno titoli sui giornali, si fa polemica, ma non si risolve il caso del detenuto. Il ministro Nordio ha ribadito che il Governo è pronto, ove richiesto dal Ministero della giustizia ungherese, a fornire ogni dettaglio relativo all'esecuzione della misura alternativa in Italia. È, cioè, falso che il ministro Nordio ed io abbiamo detto che siamo contro abbiamo manifestato tutte le nostre perplessità su una procedura che non poteva portare alla concessione degli arresti domiciliari da parte dell'autorità ungherese perché secondo noi il beneficio deve il beneficio deve essere concesso in Ungheria e poi dall'Ungheria si può cercare di avere il beneficio in Italia, compreso nell'ambasciata. L'ambasciata d'Italia in Ungheria infatti è una parte di territorio italiano quindi la responsabilità sarebbe sempre italiana. Io ho detto anche dentro l'ambasciata che non ero contrario, ma servivano tutte le cose di cui vi ho parlato perché potesse realizzarsi.

Ha inoltre spiegato il Ministro che, attraverso l'intervento del garante dei detenuti, sarà assicurata la conformità del trattamento detentivo della connazionale alle norme internazionali. Vigilerà su questo anche la Commissione europea che, per bocca della commissaria McGuinness, si è dichiarata nell'aula del Parlamento europeo disposta ad avviare una procedura di infrazione nei confronti dell'Ungheria qualora dovesse ravvisare il mancato rispetto del diritto comunitario. Ieri il nostro ambasciatore ha nuovamente incontrato la signora Salis, che gli ha sottolineato il netto miglioramento delle condizioni di detenzione; ha menzionato gli aspetti igienici (disinfestazione della cella, distribuzione di lenzuola e coperte nuove) e sanitari (riguardo sia la dieta sia la trasmissione dei referti medici richiesti), l'approccio generalmente più cortese di tutto il personale carcerario, in regime soddisfacente per quanto riguarda le comunicazioni, potendo parlare liberamente sia con la famiglia sia con l'ambasciata. La connazionale ha poi informato che le stanno dando l'accesso ai video a sostegno dell'accusa, ma non ha ancora la traduzione italiana degli atti processuali, questione che l'ambasciata tornerà a sollevare. Signor Presidente, gentili senatori, questa mia lunga ricostruzione dei fatti non è soltanto formale, ma punta a dimostrare con quanta determinazione, con quanta serietà e con quanto impegno i nostri diplomatici seguono i casi degli italiani detenuti all'estero *(Applausi)*, tutti nella stessa identica maniera, siano essi detenuti di tipo politico, siano essi detenuti non di tipo politico. Con lo stesso impegno io personalmente mi continuo a battere, per esempio, perché ci sono cittadini italiani che hanno provocato morte

Naturalmente, nei limiti che impone il rispetto del principio di sovranità giurisdizionale di un altro Stato nel proprio territorio, noi continueremo a impegnarci. A chi chiede di riportare Ilaria in Italia,

chiederei a quale soluzione stia pensando. Rispetto a quelle annunciate non ne vediamo altre. Siamo pronti ad accettare suggerimenti e proposte. L'unica per noi percorribile per un reato commesso in uno Stato membro dell'Unione è quella delle regole. Le regole europee prevedono che per chiedere gli arresti domiciliari in Italia devi prima chiederli ed ottenerli nel Paese che esercita la giurisdizione. Questa è l'idea condivisa anche dal legale ungherese, stando alle sue dichiarazioni pubblicate sulle agenzie di stampa l'altro giorno, ma, sempre a quanto riportano le agenzie, non dalla famiglia. Sono quindi due posizioni divergenti. È paradossale però che chi si erge ogni giorno a difensore dell'autonomia della magistratura chieda ora a noi di fare pressione affinché il Governo ungherese influenzi le determinazioni dei giudici. È un cortocircuito che alimenta tensioni e polemiche che danneggiano innanzitutto la causa di Ilaria. Evitiamo di trasformare una questione giudiziaria, regolata da norme nazionali ed europee ben definite, in un caso politico, che regala sicuramente titoloni sui giornali, ma non fa il bene della signora Salis. Io garantista lo sono, lo sono sempre, a prescindere dalle idee politiche di chi è coinvolto in vicende giudiziarie. Lo dimostra la mia storia politica; indipendentemente dal ruolo di Ministro degli affari esteri, ho l'onore di guidare un partito politico che del garantismo ha fatto la sua bandiera in tutte le battaglie per una giustizia equa nel nostro Paese e non solo. L'esperienza dimostra che agire con discrezione e gradualità consente di ottenere spesso i migliori risultati, proprio nell'interesse primario del detenuto. A dimostrazione di quanto ha fatto e fa ogni giorno il Governo italiano, voglio citare due casi. Il caso di Alessia Piperno, una giovane cittadina italiana, romana, appartenente alla comunità ebraica, arrestata arbitrariamente in Iran e detenuta nel carcere dei Pasdaran, colpevole soltanto di aver avuto un drone che riprendeva delle manifestazioni di giovani studenti a difesa della libertà e della democrazia in Iran. Le condizioni detentive di Alessia Piperno, cittadina di religione ebraica detenuta in Iran (guardiamo quello che sta succedendo in questi giorni), erano molto, ma molto peggiori di quelle della signora Salis. Salis. Fortunatamente però il processo non era stato incardinato, nonostante il lungo periodo di detenzione. Per questo motivo, con una lunga trattativa, il ministro Nordio ed io siamo riusciti a riportare sana e salva la giovane Alessia Piperno Con la stessa determinazione siamo riusciti a fare quello che nessun Governo era riuscito a fare prima: abbiamo ottenuto l'autorizzazione, per un giovane cittadino egiziano che aveva studiato in Italia, Patrick Zaki, a tornare dove voleva lui, cioè in Italia a studiare. Chi sostiene quindi che il Governo non si prende cura di queste vicende commette un errore. Non vale neanche il presupposto dell'appartenenza politica della signora Salis, che a me non interessa nulla, facendo io il Ministro ed essendo garantista; ne sono una dimostrazione le centinaia di dichiarazioni in vicende giudiziarie che riguardavano gli avversari politici. A me non interessa; io difendo il diritto di una persona di essere trattata in carcere con dignità. dignità. Il Governo ha fatto e continua a fare tutto ciò che è possibile per tutelare i diritti della signora Salis. Vorrei dire che non ci occupiamo soltanto della signora Salis. Ci occupiamo di tutti i cittadini italiani, nessuno escluso. Non ci sono cittadini di serie A o cittadini di serie B. Con la stessa determinazione e con lo stesso impegno con i quali si sono mossi i nostri diplomatici e il Governo, ci muoviamo per tutti gli altri italiani che sono detenuti

dubito che questa vicenda sia paragonabile agli altri casi da lei menzionati, perché qua c'è un problema di fondo, e non solo perché Ilaria Salis è stata portata al guinzaglio e legata mani e piedi all'udienza (un trattamento che viola tutta la normativa europea sui diritti della persona), oppure per le condizioni carcerarie, per gli interrogatori senza la presenza dell'avvocato e per la costrizione a firmare verbali in ungherese senza la traduzione. So che l'opinione pubblica è focalizzata su questo, ma secondo me ci sono aspetti ancora molto più inquietanti. Una giovane donna è incolpata di aver aggredito dei neonazisti: già questo stona. Una donna che picchia persone che hanno la violenza come elemento fondante della loro ideologia, poi avrebbero riportato lesioni guaribili tra i cinque e i sette giorni e non hanno neppure sporto querela: un fatto di lesioni

in Iran perché ha fatto solo questo e quest'altro, ma anche di Ilaria Salis si potrebbe dire la stessa cosa *(Applausi)*, perché un comportamento così da noi non sarebbe neanche perseguibile e men che mai si finirebbe in un carcere in custodia cautelare. Per questi fatti, la donna è da un anno in custodia cautelare in un carcere di massima sicurezza, senza neppure la prova che abbia partecipato alla rissa, ma solo per essere stata trovata in taxi con due attivisti tedeschi e aver avuto in borsa un manganello. È incolpata di appartenere alla *Hammerbande*, anche questo senza uno straccio di prova. non c'è solo un'indagine in Germania, ma la scorsa primavera, a Dresda, si è concluso un processo contro i membri della banda, accusati di diversi episodi di violenza. Nelle 800 pagine degli atti del processo il nome di Ilaria Salis I membri della banda sono stati condannati a cinque anni di carcere, non agli undici che sono stati proposti a Ilaria Salis dalla procura ungherese per un patteggiamento. Soprattutto, nelle motivazioni della sentenza tedesca si leggono concetti completamente assenti nella discussione italiana. Il giudice tedesco ha spiegato che opporsi agli estremisti di destra è un atto rispettabile ma che il monopolio dell'uso legittimo della forza appartiene allo Stato e non ai privati. Qui, invece, membri del suo Governo si scagliano contro la detenuta, sostenendo che non sia adatta a fare la maestra. ci si chiede se i neonazisti in Ungheria non godano di una tutela speciale. È già scandaloso che venga permessa la celebrazione della giornata dell'orgoglio per celebrare l'esercito hitleriano, che pare venga addirittura sostenuta con contributi pubblici, soggetti sotto tutela speciale è veramente troppo. Nessuno che provochi lesioni lievi a un'altra persona sia mai finito in un carcere di massima sicurezza, ancor meno in custodia cautelare. Mi vengono in mente le tante donne picchiate dal loro *partner*, che ovviamente non saranno così meritevoli di tutela come i neonazisti, non avendo l'Ungheria nemmeno sottoscritto la Convenzione di Istanbul. Ilaria Salis deve almeno sapere che la sua sofferenza non è vana; che mette sotto i riflettori uno Stato che non può ritenersi di diritto e che, con questa vicenda, dimostra di non essere degno di stare nell'Unione europea. Questa storia carica di fascismo e misoginia sarebbe tipica di un regime totalitario, non di una democrazia europea. Per questo, ministro Tajani, non raccontateci che l'Italia non può intromettersi nella giustizia indipendente di un altro Paese. Sappiamo tutti che la magistratura ungherese è sotto il pieno controllo di Orban e che questo è un costante fattore di diatriba con l'Unione europea. Quel Paese viola apertamente ogni principio di base di un moderno Stato di diritto, dalla proporzionalità tra comportamento illegale e pena alla presunzione di di eccezionalità di ogni misura che restringe la libertà personale prima di una condanna. Si deve alzare la voce, allora, anche nei confronti di un altro Stato. Non si può essere garantisti in Italia e sostenere che ogni Stato ha i suoi metodi, quando vengono calpestati così apertamente i diritti di una cittadina italiana.

politica e dimostra, ahimè, la tragica debolezza di questo Governo in politica estera e della sua guida della Farnesina. Abbiamo già avuto occasione di parlare della umiliazione di Roma su Expo, della Banca europea per gli investimenti e del Tribunale unificato dei brevetti.

ci dice che non è in grado di capire che ogni caso è diverso dall'altro. Vede, signor Ministro, se oggi siamo in Aula su questo caso, vuol dire che questo caso presenta delle particolarità e che non tutti i casi si possono trattare all'ammasso, come evidentemente fa la Farnesina a guida Tajani.

e non succede niente. Anche nella ricostruzione che ci ha fatto oggi del caso, ha detto che praticamente fino al 19 dicembre 2023 (la Salis è stata arrestata a febbraio del 2023, quindi per dieci mesi) la Farnesina ha

suo primo incontro, nel quale parla con il suo omologo, è del 22 gennaio. Io lo vengo a sapere il 24 gennaio, perché rispondete a una mia interrogazione. Quindi, il caso non è esploso dopo, perché questo Parlamento si era già interessato a Ilaria Salis. Lei il 24 gennaio mi dice che lei, il 22 gennaio, ha incontrato il Ministro suo omologo. Poi oggi ci ha detto che il 30 gennaio, la nostra Presidente del Consiglio ha parlato con Orban. Mi dite che sono stati dati consigli giuridici da parte del ministro Nordio, sempre in questi giorni, ma io le chiedo: dall'11 Febbraio 2023 fino a dicembre che cosa avete fatto? Adesso lei dice che bisogna tenere la cosa sotto silenzio, perché è più facile operare quando siamo sotto silenzio, ma questo caso è stato sotto silenzio fino al mese di ottobre. Voi avete avuto tempo da febbraio a ottobre di agire in modo silenziosissimo e non avete fatto nulla. *(Applausi)*. lei dice che non riconoscevamo la giurisdizione, ma poi è venuto qui a dirci che gli arresti domiciliari a Salis non si possono dare nell'ambasciata italiana per tutte altre ragioni. Ha detto che l'ambasciata non è attrezzata, però se era attrezzata per i marò, può essere attrezzata anche per la Salis, mi perdoni, anche se i casi sono giuridicamente diversi. Lei ha giustificato la questione di non poter dare i domiciliari alla Salis nell'ambasciata per una questione logistica, se ho capito bene. Allora il problema sa qual è? è? Qui siamo davanti a una pesantissima incompetenza, perché è vero che vi siete svegliati (adesso parlate con Orban e con il Ministro), ma l'avete fatto da quando l'opinione pubblica è stata colpita. Prima che cosa è successo? Niente. Oppure, c'è un'altra possibilità, un'altra possibilità, cioè che il Governo in questione, il Governo Orban, con il quale si va a fare la parata di Dio, Patria e famiglia, è il Governo di un partito che promette di entrare nel Gruppo presieduto dalla Presidente del Consiglio. Allora, viene legittimo il sospetto che se non c'è incompetenza - e io mi auguro che sia così - ci sia della malafede, perché vuol dire che voi quantomeno non avete utilizzato i vostri buoni uffici e i rapporti politici che avete con Fidesz, il partito di Orban, per chiedere a Orban una cosa che può fare. Come diceva la collega Unterberger, l'indipendenza della magistratura in Ungheria non esiste: è un argomento puramente formale, altrimenti non agiremmo nei confronti del dell'Ungheria con gli strumenti dei trattati Concluda per favore. aveste parlato con i vostri omologhi nel mese di luglio o nel mese di marzo, sapendo che una nostra connazionale era praticamente al 41-*bis*, probabilmente la situazione sarebbe stata già risolta. Quindi, o siete incompetenti, o siete in malafede. *(Applausi)*. *(Misto-AVS)*. Signor Ministro, devo dire che fino a stamattina ero molto arrabbiata. Adesso sono molto avvilita dopo averla ascoltata. Non voglio ripetere quello che hanno già sottolineato i miei colleghi che mi hanno preceduta, però voglio ricordare

"profondo dolore e sorpresa" nel vedere Ilaria Salis ammanettata in udienza, quindi come a far capire di non sapere nulla di tutto questo. In realtà, oltre all'elenco delle cose fatte che ci ha appena letto, letto, lei e tutti i suoi colleghi, compresa la presidente Meloni, eravate al corrente da subito di quello che accadeva, perché il 22 marzo 2023 era stata scritta una lettera via PEC da parte della famiglia di Ilaria alla Presidente del Consiglio,

Ilaria Salis, lei ha fatto queste dichiarazioni e il ministro Nordio dà addirittura consigli: il consiglio del nostro Ministro ai familiari di Ilaria Salis è di prendere i domiciliari in Ungheria. Ma lei è al corrente del fatto che i presunti picchiati da parte di Ilaria - dobbiamo infatti usare ancora

Questo è quello che siete in grado di fare? Per quanto riguarda il caos mediatico, ho appena ribadito che il vero caso è esploso esattamente il 10 gennaio, in seguito alla mia conferenza stampa. Avete avuto un anno di tempo, potevate fare di tutto e oggi lamentate che il

Ministro, che l'Ungheria imponga alla cittadina italiana Ilaria Salis condizioni di detenzione del tutto inumane e degradanti è ormai impossibile negarlo: l'abbiamo vista tutti in catene il giorno dell'udienza; non si poteva più negare, ormai il danno era fatto. Come prima cosa chiediamo come sia possibile che ad oggi non sia stata inviata una formale ed ufficiale protesta per la grave violazione dei diritti umani e civili subiti da Ilaria Salis. Quello che è più grave però e che è del tutto inaccettabile è il fatto che siano rimaste inascoltate per ben un anno tutte le documentate richieste di aiuto della donna e della famiglia. Trovo gravissimo che, innanzi a quelle foto, la Presidente del Consiglio si sia limitata a dire che si augura che Ilaria Salis sia innocente e riesca a dimostrare la propria innocenza, incurante del più fondamentale dei principi del diritto penale, ossia la presunzione di innocenza. Ilaria

Trovo gravissimo che il ministro Nordio dinanzi a quelle foto si sia mostrato sorpreso. Com'è possibile mostrarsi sorpresi il 19 gennaio, quando è datata a quasi quattro mesi prima, il 2 ottobre 2023, la lettera che Ilaria ha spedito al consolato in Ungheria in cui descrive con dovizia di particolari le condizioni di detenzione impostele da Budapest? Il 10 gennaio è stato lanciato l'appello. Quindi diciamo che è stato trattato tutto con la dovuta urgenza? Diciamo che vi siete attivati? Direi che a questo punto possiamo anche avere l'accesso agli atti, com'è nostro diritto, e - cosa che abbiamo fatto questa mattina, come Alleanza Verdi e Sinistra - chiediamo l'invio di una richiesta ufficiale

Signor Presidente, innanzitutto vogliamo ringraziare il Ministro degli affari esteri e Vice *Premier*, che è venuto prontamente a rispondere in Parlamento sul caso Salis,

le proprie scuse per quanto accaduto nel dibattito pubblico nei giorni passati; invece ho sentito cose fuori dal mondo, come affermazioni riportate ed applaudite da una parte dell'Assemblea,

tant'è, questi sono i giorni che passiamo. Il suo appello a fare in modo che gli interessi di Ilaria Salis avessero la precedenza mi sembra che non sia stato colto e non sia stato assolutamente sostenuto. La polemica politica rischierà di penalizzare questa situazione, come lei ha detto puntualmente. La sua informativa, infatti, è stata puntualissima e chiarissima e rende merito a un lavoro fatto ben prima delle polemiche di questi giorni che, alla luce delle sue dichiarazioni, si rivelano totalmente infondate e fuori luogo. Spero che qualcuno possa davvero comprenderlo ed evitare gli atteggiamenti a cui abbiamo assistito, anche perché le prediche a cui abbiamo assistito

in Ungheria e in Italia e tutti i rappresentanti della Farnesina, per essersi adoperati fin dal primo minuto, com'è stato ben riportato, di questa purtroppo triste vicenda. io ricordare che non ho visto questo slancio internazionale da parte della sinistra e dei Governi di sinistra quando altri Paesi europei davano riparo a brigatisti e terroristi con pesanti condanne nel nostro Paese, di fronte al silenzio di una parte politica che non ha mai chiesto che ci fossero davvero provvedimenti conseguenti alle richieste dell'Italia. come abbiamo saputo dalle dichiarazioni del signor Ministro, sono addirittura 2.405 gli italiani in stato di detenzione all'estero e siamo confortati dal fatto che, come lei ha opportunamente detto, noi non lasciamo nessuno da solo, sarebbe spiacevole. Io ho sentito dichiarazioni, ma non credo che la Farnesina debba entrare nel merito dei processi e dei procedimenti. È chiaro che vanno analizzate anche le situazioni, ma noi rifiutiamo l'idea che ci siano italiani detenuti all'estero di serie A e di serie B; gli italiani detenuti all'estero devono essere seguiti come voi ben fate e come contiamo che questo Governo

che liberare un detenuto all'estero non è compito del Governo italiano, non può esserlo; il compito del Governo, come ha già fatto, è quello di ribadire che va rispettato il diritto di ogni detenuto. Ha fatto bene a convocare l'ambasciatore ungherese a Roma, perché è stato un atto politico forte per esprimere questa posizione. Non si può che biasimare, infatti - l'ha già fatto con chiarezza lei, ma l'abbiamo fatto tutti con dichiarazioni pubbliche molto chiare - il modo in cui Ilaria Salis è stata tradotta in aula, non rispettoso degli elementari diritti alla dignità. I diritti di un cittadino in stato di detenzione devono essere rispettati sia in carcere sia in un'aula di tribunale. Bene che la *premier* Giorgia Meloni, come lei ha detto, abbia incontrato il ministro ungherese Viktor Orban su questo tema. Vanno anche ricordate - l'ha ricordato lei e glie ne va dato merito - le vicende di Alessia Piperno e di Patrick Zaki. Fortuna che qualcuno se n'è occupato in modo adeguato, perché probabilmente in altre situazioni sarebbero ancora dove non dovevano essere. Anche in questo caso, però, il Governo sta agendo nell'interesse della cittadina italiana Salis ed è bene che si sia data anche la propria disponibilità, qualora vengano concessi gli arresti domiciliari in Ungheria, a mettere a disposizione un luogo adeguato. È chiaro, tuttavia, che spetta all'autorità giudiziaria ungherese e in base a una richiesta dell'avvocato, che chiaramente dev'essere fatta - speriamo che venga fatta - concedere gli arresti domiciliari in Ungheria e poi bisognerà lavorare perché questi arresti domiciliari possano essere tradotti in arresti domiciliari nel nostro Paese. Noi comprendiamo lo stato d'animo del padre di Ilaria Salis, ma non possiamo condividere le sue dichiarazioni, mentre ci sentiamo di condividere e di sostenere pienamente le iniziative italiane che il Governo ha messo in campo per chiedere il rispetto del diritto europeo sullo stato di detenzione e sul rispetto della persona.

allora parliamo veramente di una storia straordinaria e terribile nella sua straordinarietà. Un anno trascorso nel silenzio delle istituzioni, signor Ministro, checché se ne dica, silenzio che non deriva dalla necessità di mantenere riservate certe notizie, perché magari nel frattempo ci si adoperava per garantire condizioni detentive dignitose a Ilaria Salis o magari per farla rientrare nel suo Paese. Questo silenzio, signor Ministro, deriva dall'assoluta mancata conoscenza di ciò che Ilaria stava vivendo, nonostante la famiglia e lei stessa, fin da subito si fossero adoperate per far conoscere quello che stava stava vivendo. Dobbiamo immaginare la sua paura e la rabbia della famiglia e degli amici di Ilaria. Immaginiamo il senso di solitudine e di abbandono vissuto da questa ragazza, nostra concittadina, arrestata - ripetiamolo - un anno fa, in un Paese della "civilissima" Europa, la cui condizione detentiva non è assolutamente dignitosa, né rispettosa della dignità della persona. Questo non è mai accettabile, figuriamoci se può esserlo in un Paese con il quale il nostro *Premier* non perde occasione per rimarcare e difendere il rapporto amichevole con il presidente Orban, il quale a sua volta ha dichiarato di avere con Giorgia Meloni una visione comune del mondo. Signor Presidente, questo sicuramente per noi non è assolutamente rassicurante. Come cittadina italiana e come parlamentare, sento di dover chiedere scusa ad Ilaria per quanto è successo. Sento però, Ministro, che lei avrebbe dovuto farlo prima di tutti noi, ammettendo di aver lasciato sola Ilaria per troppo tempo, senza quel sostegno e quell'incoraggiamento che - mi creda - chi vive quella condizione necessita come l'aria che lei respira, signor Ministro. Ora bisogna recuperare, bisogna stare vicino ad Ilaria, è necessario che le arrivino tutta la nostra vicinanza e l'impegno che tornerà a casa. Il ministro Nordio ha dichiarato che l'Italia non è un Paese affidabile per l'estradizione dei nostri connazionali detenuti all'estero. Purtroppo è la verità. Lo so bene, però lei può impegnarsi per invertire questa tendenza. Dico lo so bene, perché, signor Ministro, sono un'amica di Enrico Forti. So che il Governo si sta occupando della storia di Chico. Conosco Chico dal 2011 e tutti i Governi che si sono succeduti si sono occupati di lui. Tutti i Governi hanno fatto piccoli passi in avanti. È complicato, e lo sappiamo. Tra l'altro, oggi è il compleanno di Chico Forti, il ventiquattresimo che che trascorre in un carcere di massima sicurezza in Florida e, mi permetta, Presidente di rivolgergli anche da qui gli auguri di buon compleanno. Quindi, sintetizzando, perché questo è il messaggio a nostro avviso più importante: è davvero fondamentale, determinante non abbandonare, non trascurare - questo forse è il termine più adatto - i nostri concittadini detenuti all'estero e far sentire loro l'interesse, la vicinanza delle istituzioni. Signor Ministro, smentisca il ministro Nordio.

Aula e per il supporto a tutti quei cittadini italiani detenuti all'estero che, avendo avuto appunto problemi con la giustizia, si trovano in carcere, magari in realtà dove i requisiti minimi per il rispetto e la tutela dei diritti umani vengono meno. Questo supporto avviene proprio attraverso il suo Ministero, la Farnesina, e le nostre ambasciate. Grazie anche al lavoro della Commissione per i diritti umani, che ho avuto ho tuttora l'onore di presiedere. Nel novembre del 2019 la Farnesina ha pubblicato un prezioso *vademecum* proprio per far sì che i detenuti all'estero e i loro familiari avessero avessero un supporto per tutte le iniziative che possono aiutarli in una situazione di disagio. La guida messa a punto è stata concepita come uno strumento di facile consultazione, un ausilio per le persone che si trovano in maggiore difficoltà a causa della non conoscenza della lingua e del diritto locale e spesso con l'impossibilità di ricevere medicinali, oltre che con i familiari distanti. Nel *vademecum* viene illustrato cosa fa e cosa non può fare la rappresentanza diplomatica e contiene la guida nelle pratiche per l'estradizione. Per entrare nel merito specifico del caso di Ilaria Salis, vorrei

L'ambasciata viene informata il 13 febbraio in tarda serata. Il giorno dopo, nonostante lo strettissimo tempo a disposizione, l'addetto consolare che parla la lingua ungherese riesce a partecipare all'udienza con il gip, dove riesce ad avere il primo incontro con Ilaria. Il 15, cioè un giorno dopo questo incontro, l'addetto informa la famiglia sul colloquio avuto con la figlia e su una serie di questioni circa l'invio di beni personali, le modalità di visita e le azioni che l'ambasciata avrebbe messo in atto per assisterla. La difficoltà riscontrata nel mettere in contatto Ilaria con la propria famiglia sta nel fatto che, nella fase delle indagini, le autorità ungheresi hanno vietato i contatti con la famiglia; difficoltà riscontrata anche per la richiesta di visita consolare autorizzata dopo circa un mese dalla richiesta iniziale.

alle visite e alle telefonate che, infatti, con il tempo si sono fatte più frequenti. Oggi Ilaria può telefonare liberamente all'ambasciata e ricevere visite. Sicuramente le immagini di lei tradotta in aula con i ceppi ai piedi e trattenuta con una catena non si possono guardare e non si possono accettare.

ci sono oltre 2.400 detenuti italiani nel mondo, spesso in condizioni in cui il rispetto della dignità umana è lontano da poter essere definito come tale,

Il Governo interverrà con ogni strumento a disposizione nei casi in cui vi siano violazioni nei confronti dei nostri connazionali, tenendo conto del limite della sovranità giurisdizionale. È un lavoro costante quello che spesso viene fatto - come è stato anche dimostrato nel caso di Ilaria Salis sottotraccia proprio perché a volte la sovraesposizione crea un danno anziché dare un contributo di aiuto alla persona in difficoltà. Fare del caso Salis un caso politico, come è diventato, non fa il bene della ragazza e - come è stato confermato da più parti - la necessità di mantenere i toni bassi, proprio per non far irrigidire la controparte e non vanificare il lavoro che l'ambasciata ha fatto fino ad oggi, sembra essere caduto nel vuoto. Ilaria Salis non può essere utilizzata come strumento elettorale per colpire Orban o il Governo italiano *(Applausi),* e non si può far leva su quella che è l'emotività della famiglia che in questo momento sta soffrendo. Se realmente quello a cui si vuole arrivare è il rispetto delle regole umanitarie ed europeo, oltre che un giusto processo, la via non è quella dei *flashmob*, della spettacolarizzazione politica, ma è quella del senso di responsabilità di ognuno di noi.

Non vorrei che passasse il concetto - come si è appena sentito in quest'Aula - che la violenza è da condannare solamente quando la persona che la subisce è di destra. *(Applausi)*. Ecco, questo è un concetto che sinceramente vorrei che in questa Aula non fosse applaudito, perché la violenza va combattuta senza se e senza ma. *(Applausi)*.

il Gruppo Partito Democratico e la comunità democratica condannano ogni tipo di violenza, al di là di qualsiasi colore politico, sempre e dovunque, e pensano che tutti i cittadini italiani ed europei

tanti incarichi (Presidente del Parlamento europeo e Commissario europeo), da non sapere che questo è un caso simbolico. Il Ministro degli affari esteri italiano non può permettersi di paragonare situazioni dell'Iran e dell'Egitto a una situazione che è nel cuore dell'Europa, della civile Europa, in Ungheria. I diritti in Ungheria, in Italia, in Francia e in Germania devono essere rispettati e tutelati nella stessa maniera. Questo è il punto centrale, cui ci ha richiamato anche la commissaria europea McGuinness, che ha dato una valutazione diversa dalla vostra rispetto alla decisione quadro 829 Lo dico perché stiamo parlando di un tema centrale che è la vera posta in gioco. Oggi non parliamo del caso di Ilaria Salis dal punto di vista giudiziario, su cui ci sarà un processo e potremo poi esprimerci ognuno con le sue valutazioni. Oggi la posta in gioco è lo Stato di diritto all'interno dell'Unione europea che viene messo in discussione dall'Ungheria. Io non vorrei che ci assuefacessimo ormai all'idea che Orban può dire tutto e il contrario di tutto impunito. Siccome lei stesso ha partecipato alle decisioni che hanno bloccato i fondi all'Ungheria, proprio sul tema delle libertà fondamentali e della separazione dei poteri, e ha votato anche lei a favore del blocco di quei fondi, fa sorridere pensare e sentire Ministri di questo Governo che si appellano all'indipendenza della magistratura in Ungheria, quando sa benissimo che è merce di scambio ogni decisione da parte di Orban. *(Applausi)*. Qualsiasi cosa: l'entrata nella NATO della Svezia la decisione di prendere e definire un testo unico su Israele e Hamas. Minacciano ormai il veto ovunque e ogni cosa è occasione di negoziato con loro. Siete stati bravi in Egitto e siete stati bravi in Iran. Dovrebbe essere molto più facile ottenere un risultato in Europa, tra l'altro con un vostro alleato e amico della presidente Meloni, che si accinge a entrare nel Gruppo dei conservatori europei. risposto il Governo davanti ai continui richiami e alle lettere che sono arrivate (il 23 marzo scorso è passato più di un anno dalla prima lettera del padre di Ilaria Salis, che ha riscritto in autunno). che ha riscritto in autunno). Il Governo non ha risposto. I primi incontri ci sono stati alla fine di gennaio, quando il primo dicembre il Partito Democratico ha interrogato questo Governo per sapere cosa intendesse fare nei confronti dell'Ungheria. Noi stiamo ancora aspettando una risposta a quell'interrogazione. *(Applausi)*. Mi chiedo, quando ai primi di dicembre Cuno Tarfusser, che non è uno qualunque, ma è stato vice presidente della Corte penale internazionale e sostituto procuratore della corte d'appello di Milano, chiede di non estradare Gabriele Marchesi, accusato degli stessi reati della Salis, e indica anche la lettera del padre della Salis a questo Governo, in cui si scriveva anche "legata, ammanettata e portata con un guinzaglio" - quindi tutto ciò lo si sapeva in autunno e lo si sapeva a dicembre noi ci chiediamo che cosa ha fatto il Governo in quest'anno. Perché ha dovuto aspettare gennaio? Questo è il punto chiave. *(Applausi)*. A me rassicura tutto l'elenco dei punti che sono stati fatti

non mi rassicura che il Governo italiano abbia dovuto aspettare la fine di gennaio per incontrare il Ministro della giustizia ungherese. Questo è il punto centrale. Cosa ha fatto il Governo in tutti questi mesi? Per questo motivo abbiamo sollevato un caso. Mi sembra abbastanza evidente che questo è il punto centrale. Chiudo su un punto, che è il tema dello Stato di diritto all'interno dell'Unione europea. Questo è il punto fondamentale che viene oggi messo in discussione con un trattamento lesivo dei più elementari diritti umani - un collega diceva prima che è peggio del 41-*bis* in Italia per un reato che poi dovrà essere accertato e che è molto meno grave rispetto ai reati per cui si viene colpiti con quella sanzione. Allora io mi chiedo e lo chiedo soprattutto ai patrioti,

francesi o i tedeschi - la reazione del Governo in questi mesi qual è stata? I patrioti danno l'idea di aver abbandonato questa bandiera, la bandiera della difesa dell'italianità. Perché lo hanno fatto? Lo hanno fatto forse perché Orban, in compagnia di Zemmour, quel signore che ha fatto campagna elettorale denunciando l'idea di parità di genere ed evocando una battaglia per annettere addirittura le Regioni del Nord Italia alla Francia - questo ha fatto - è entrato l'altro giorno all'interno del Gruppo guidato dalla Presidente del Consiglio italiana? Patrioti, dove siete? Battete un colpo.

ringraziare il ministro Tajani per la sua precisa e puntuale informativa che ha voluto fare oggi in quest'Aula. Non avevamo dubbi, Ministro, lo avevamo già anticipato nel dibattito che c'è stato la scorsa settimana; mi riferisco all'interessamento che il Governo ha posto su questa vicenda sin da subito. Mi piace ricordare da dove lei è partito, ricordando cioè come l'Italia sia la Patria del diritto, la culla di Cesare Beccaria, il luogo dove la dignità umana è sempre stata salvaguardata, sottolineata e tutelata proprio in quanto italiani e proprio in quanto culla di una civiltà che, sinceramente, non fa sconti a nessuno. Lo dico perché il suo interesse, l'interesse di questo Governo, è per tutti i detenuti italiani all'estero - come è stato anche qui ricordato - e non riguarda solo la vicenda di Ilaria Salis.

echi terribili in quest'Aula, quando qualcuno ha parlato di giustificazione della violenza nei confronti di persone che la pensano diversamente da altre, che poi sono giustificate a usare quella violenza. E purtroppo vi sono stati applausi anche da parte del Gruppo Partito che non funziona, perché allora si chiarisce il perché siamo qui. Noi siamo qui per cercare una soluzione per il caso Salis o siamo qui per fare polemica politica? Noi dovremmo Noi dovremmo rispettare, solamente e semplicemente, non tanto quello che dice il ministro Tajani, il Presidente del Consiglio e tantomeno quello che dico io, ma quello che dice il padre di Ilaria Salis. Il padre di mettere a tacere la situazione, di non creare un caso politico su questa vicenda, perché ciò non aiuta. E non lo dice adesso. Io non voglio ora rifare l'elenco di tutti gli interventi che il ministro Tajani ha riportato all'inizio di questa informativa. Ma, se dobbiamo parlare, e non in malafede - certe volte la vedo arrivare da altri banchi - dobbiamo ricordare quello che ci ha detto il Ministro. Poi, se uno viene qui con gli interventi prestampati, perché servono a fare un comunicato stampa, va bene qualunque cosa; ma il Ministro ci ha detto che, dal 15 febbraio dello scorso anno, l'ambasciata italiana e quindi il Ministero degli Esteri, si sono attivati in una serie di interventi. Sono intervenuti a inizio febbraio, a metà febbraio, a fine febbraio, a marzo, ad aprile, a maggio, a luglio. Come si fa a dire che il Governo italiano non è intervenuto? Siamo in malafede, cari colleghi. Siamo davvero in malafede! *(Applausi)*. che cosa volete che si faccia in più, rispetto a quello che è stato fatto? È stato convocato l'ambasciatore ungherese: neanche in tempo di guerra si prende questa

Ora, voi potete dire che quello ungherese è un popolo di nazisti, di terribili razzisti. Dite quello che volete, ma c'è un processo democratico chiaro. E non si può essere democratici solo quando vince la parte che si ha in simpatia, perché questa è un'altra storia. sul tema dell'autonomia della magistratura all'interno dello Stato ungherese, al di sopra vi è l'Unione europea, con tutto quello che sappiamo. tutto da verificare; ma, fino a quel momento, la magistratura ungherese è l'unica magistratura che può decidere le sorti della nostra connazionale, sulla quale il Governo ha fatto tutto quello che era possibile fare.

perché c'è stato un lavoro attento, attivo, diplomatico, senza cercare titoli di giornali, comunicati stampa e altre attenzioni, che in questo caso, forse, fanno appunto davvero alla malafede. Noi lavoriamo così. E siamo sicuri che, grazie all'intervento del Governo, anche questa situazione avrà il risultato che deve avere.

vorrei ribadire al presidente La Russa, attraverso lei - e mi auguro che il presidente Malan convenga su questo - che ancora una volta ci sono colleghe e colleghi che sono stati penalizzati dalla testardaggine di alcuni Presidenti di Commissione. Avevamo chiesto di evitare, durante questi lavori, di convocare l'Ufficio di Presidenza della Commissione affari costituzionali, perché avevamo bisogno - come lei sa - di definire prima un percorso, e in ogni caso dovevamo consentire a tutti i colleghi di seguire l'informativa del ministro Tajani. Ma la cosa che ci lascia interdetti è che questa sensibilità e questa attenzione non sono state tenute in considerazione nemmeno nelle Commissioni congiunte. o era qui o era lì; e, siccome era qui, perché interveniva in Aula per conto del Partito democratico, non poteva essere lì. E intanto in quella sede i lavori vanno avanti. Lo dico, presidente Ronzulli, perché è evidente che anche il dibattito di questa mattina non ha sortito effetti e noi davvero chiediamo una convocazione della Conferenza dei Capigruppo prima di incominciare i lavori la settimana prossima. Non siamo in grado di garantire, almeno da parte nostra, lo svolgimento dei lavori di un calendario che è già saltato. Infatti, come lei sa, perché ha partecipato all'ultima Conferenza dei Capigruppo, noi ci ritroviamo in questo momento con il disegno di legge Nordio ancora aperto, con emendamenti da votare e con probabile voto finale. Ci ritroviamo la legge di delegazione europea con la discussione generale fatta, ma non sappiamo se possiamo affrontarla prima dell'ossessivo provvedimento su Italia-Albania che, non per volontà dell'Assemblea, ma per il Governo che spinge, dovrebbe superare tutti gli altri, ma in realtà in Commissione non abbiamo ancora iniziato a trattare gli emendamenti. Il disegno di legge sul cyberbullismo è stato accantonato, e non si sa in quale angolo dei nostri lavori sia finito. ovviamente le opposizioni stanno aspettando il ministro Fitto da sei mesi, perché sull'affare assegnato è scomparso. Non sappiamo dove sia finito. La Commissione affari europei chiede la sua presenza da sei mesi e noi non siamo più in grado, perché son saltate le regole - lo dico al presidente Malan - e sono saltati anche i criteri minimi di rispetto della nostra convivenza in quest'Aula e nelle Commissioni.

d'onore. Nell'altro ramo del Parlamento non ha funzionato molto bene e qui, se ci organizziamo, forse riusciamo a farlo funzionare; certo, diventerebbe molto complicato tradurre il presidente Balboni, un esercizio che possono fare i suoi compagni di partito. Le chiedo, pertanto, Presidente, di chiedere al presidente La Russa di ricominciare da una al presidente La Russa di ricominciare da una Conferenza dei Capigruppo. Noi non siamo nella condizione di iniziare la prossima settimana, e non a causa nostra, ma a causa del caos che si è creato per evidenti forzature del Governo sull'intera Aula e della maggioranza, che evidentemente non è nemmeno compatta sulla definizione delle priorità. ora non è più rappresentato e non abbia la voglia spasmodica di ripartire da Italia-Albania.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 con il *question time*. *(La seduta, sospesa

al Ministro della difesa, evidenzio in premessa che il mar Rosso è, in relazione alle comunicazioni via mare, uno snodo cruciale per il commercio mondiale; dopo gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre scorso e l'inizio delle operazioni israeliane nella striscia di Gaza, i ribelli yemeniti di Ansar Allah, sostenuti dall'Iran, hanno perpetrato ripetuti attacchi contro le navi in transito nel mar Rosso, in particolare nello stretto di Bab el-Mandeb, mettendo a rischio la libertà e la sicurezza della navigazione lungo una delle rotte commerciali più importanti al mondo e arrecando danno alle compagnie di navigazione. Questi attacchi hanno indotto molte compagnie di navigazione a rinunciare all'ingresso nel Mediterraneo, attraverso il canale di Suez, e a circumnavigare l'Africa; le deviazioni stanno comportando un impatto enorme sia sui tempi di navigazione, sia sui costi del trasporto delle merci, aumentati anche a causa dei maggiori costi assicurativi conseguenti all'elevato rischio di attacchi. La crisi rischia così di ridurre l'importanza commerciale dei principali porti italiani, inficiando la centralità del Mediterraneo nella rotta commerciale che collega l'Asia all'Europa e agli Stati Uniti. Lo scorso dicembre, al fine di contrastare gli attacchi e le minacce dei ribelli yemeniti di Ansar Allah, il Segretario alla difesa Austin, ha annunciato l'avvio dell'operazione Prosperity guardian, di natura difensiva, imperniata su una coalizione multinazionale ed inserita nella Combined Task Force 153, una delle cinque *task force* multinazionali che compongono le *combined maritime force* (CMF). Nella notte tra l'11 e il 12 gennaio 2024, a causa del perdurare degli attacchi, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, con il supporto non operativo di Paesi Bassi, Bahrein, Nuova Zelanda, Canada, Australia, Danimarca, Germania e Corea del Sud, hanno avviato una serie di attacchi contro le posizioni Houthi sul territorio yemenita, con lo scopo di degradarne le capacità operative. Lo scorso 22 gennaio si è tenuta a Bruxelles la riunione del Consiglio affari esteri dell'Unione europea, in cui è stata discussa la situazione nel mar Rosso ed è stato raggiunto un accordo di principio sull'avvio di una nuova missione militare UE a protezione delle navi commerciali che attraversano l'area. Tale missione incrementerebbe di fatto la presenza italiana e alleata nell'area: l'Italia, in particolare, è già presente con nave Martinengo, posizionata a Nord di Bab el-Mandeb, che ha da poco avvicendato nave Fasan; inoltre, l'Italia partecipa altresì all'operazione Atalanta, una missione navale europea di cui il nostro Paese assumerà a breve il comando, attiva attiva dal 2008 al largo della Somalia con l'obiettivo di contrastare le attività di pirateria. È del 4 febbraio la notizia che il comando tattico, ovvero la responsabilità della condotta in mare delle attività rientranti (denominata Aspides, «scudo» in greco), sarà assegnato all'Italia. Si chiede di sapere quali siano le iniziative in atto nell'area del mar Rosso a tutela del traffico mercantile, in transito per lo stretto di Bab Bab el-Mandeb e per il canale di Suez, e in particolare quali siano la natura e gli obiettivi della nuova missione e se essa preveda il coinvolgimento di altri Paesi. *(Applausi)*.

ringrazio la senatrice Mieli perché mi fornisce l'opportunità di fare il punto anche in questa sede sui recenti sviluppi della situazione nel mar Rosso, nel golfo di Aden e sulle decisioni assunte in sede europea in relazione all'imminente invio di una missione navale in un'area cruciale per il commercio e l'economia globale. Gli attacchi Houthi hanno determinato sin da subito un serio pericolo per chi opera in mare, inducendo le principali imprese di navigazione e compagnie marittime a evitare il transito nello stretto di Bab el-Mandeb e di conseguenza da Suez, optando per la circumnavigazione del Capo di Buona Speranza. Non passare da Suez porta a un aumento dei tempi di navigazione di dieci, dodici giorni, a un deciso incremento di costi di trasporto - in alcuni casi quintuplicati alla marginalizzazione dei porti del Mediterraneo, con un ulteriore impatto negativo sull'economia europea e italiana in particolare. Le navi russe o cinesi non vengono attaccate dagli ciò crea uno svantaggio competitivo e altera le regole del libero mercato, generando una minaccia alla sicurezza della navigazione e alla nostra stabilità economica. Quello in atto è quindi un vero e proprio

le sue merci con loro viaggeranno in modo sicuro e non saranno attaccate, offrendo un vantaggio commerciale in più rispetto a quello che potevano fornire i concorrenti europei e americani. Come sapete, l'Italia fin da subito ha ritenuto di agire per ripristinare la sicurezza e la libertà di navigazione nell'area, inviando un'unità navale, la fregata Fasan, oggi sostituita con nave Martinengo, con compiti di *maritime situational awareness* e di autodifesa estesa a favore del naviglio in transito sul mar Rosso. Al contempo, in sinergia con gli Esteri, abbiamo stimolato e supportato il rapido avvio di un'iniziativa dell'Unione europea, poi denominata Aspides. Con Parigi e Berlino in particolare, stiamo fortemente supportando il lancio di questa operazione che dovrebbe agire nel mar Rosso parte del Golfo Persico, inglobando l'altra operazione europea Emasoh, finalizzata alla sorveglianza dello Stato di Hormuz, delle cui strutture, capacità e competenze potrà avvalersi, a tutto vantaggio della rapidità decisionale ed esecutiva. Le navi militari europee svolgeranno compiti di protezione e scorta del naviglio e supporto di *maritime situational awareness*, mantenendo uno stretto coordinamento con Atlanta, che ha preminenti compiti antipirateria, con cui Aspides condividerà parte dell'area operazioni, e con Prosperity guardian, missione a carattere difensivo che - come ricordava la senatrice interrogante - è imperniata su una coalizione multinazionale inserita nella Combined task force 153. Aspides è una missione difensiva dell'Unione europea, che auspichiamo possa prevedere la partecipazione di altri Paesi extraeuropei. Gli assetti europei di previsto impiego per l'operazione comprenderanno un minimo di tre unità navali, supporto *intelligence* e logistico, capacità di sorveglianza e di *early warning* aereo; protezione *cyber*, supporto satellitare, comunicazione strategica. Oltre al fondamentale contributo in termini di assetti navali, stiamo valutando la possibilità di fornire assetti aerei con capacità di sorveglianza. Anche in ragione delle nostre riconosciute capacità, l'Unione europea ha chiesto all'Italia di fornire il Force commander dell'operazione. In sostanza, fintanto che permarrà l'attuale situazione crisi, l'Italia manterrà permanentemente almeno un'unità navale nazionale nel mar Rosso e supporterà in maniera diretta o indiretta le operazioni che abbiano il mandato di tutelare la sicurezza e il diritto internazionale. Quando il processo decisionale sarà concluso, presumibilmente con la riunione dei ministri degli esteri del prossimo 19 febbraio, la Difesa predisporrà i dettagli necessari e potrà valutare più compiutamente quale contributo operativo fornire, inserendo nella delibera della missione 2024 per la prevista autorizzazione parlamentare, il nuovo dispositivo; un passaggio - voglio rassicurare tutti - al quale non intendiamo derogare. Al riguardo, il quadro in divenire prefigura tuttavia un accresciuto impiego della difesa non preventivabile in fase di predisposizione delle assegnazioni finanziarie per gli impegni 2024 che - lo dico fin d'ora, e non sapevo di essere seduto di fianco al ministro Giorgetti, ma, lo ammetto difficilmente sarà compensabile con una revisione in senso riduttivo degli altri impegni nelle ulteriori aree di crisi che ci vedono impegnati. Ritengo dunque che il nostro impegno per la sicurezza del mar Rosso debba trovare ristoro tramite finanziamenti aggiuntivi che vadano oltre il periodo previsto con la recente approvazione della legge di bilancio. conclusione, onorevoli senatori, la gravità della situazione e delle potenziali conseguenze impongono di agire con urgenza ed efficacia insieme ai nostri alleati per ripristinare il diritto internazionale e il libero transito delle merci. Questo è ciò che stiamo facendo e che abbiamo chiesto di fare all'Unione europea con una missione di difesa e non di offesa.

ci stiamo, vi state facendo carico per la protezione dei traffici nel mar Rosso, testimonia - e di questo siamo più che certi - l'impegno del suo Dicastero per la sicurezza della navigazione in un'area fondamentale, oltre che per l'economia globale, anche per i nostri stessi interessi nazionali. Nel ringraziare lei, voglio ringraziare la Marina militare e tutte le nostre Forze armate *(Applausi)* per la credibilità che, con il loro operato, conferiscono sempre più all'Italia.

gioca un ruolo cruciale nelle politiche economiche quando si intende migliorare l'efficienza del settore pubblico. Qualche mese fa abbiamo approvato la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e, come obiettivo di politica economica, ci siamo posti un piano di dismissioni di *asset* non strategici per un valore pari all'1 per cento del prodotto interno lordo. Le privatizzazioni servono al nostro Paese, servono per crescere, servono alla competitività e all'efficienza del settore pubblico. Come dicevo, tralasciando gli *asset* strategici, dove invece lo Stato deve giocare sempre un ruolo più importante, parliamo di *asset* non strategici e, quindi, di settori del servizio pubblico quali possono essere i servizi portuali, il trasporto pubblico, la valorizzazione anche dei rifiuti e il loro smaltimento, all'interno

all'interno delle quali bisogna poi trovare questa sinergia tra pubblico e privato, serve attrarre questi investimenti. Lei, Ministro, sa benissimo che questo valore è oggi un valore di risorse economiche importanti che lo Stato può risparmiare. L'uno per cento del prodotto interno lordo oggi del nostro Paese vale 20 miliardi di euro di risparmio nel triennio 2024-2026. Ribadendo che sugli *asset* strategici invece deve essere forte la presenza dello Stato, noi dobbiamo intendere queste dismissioni non come un buttare via cose che non servono più al nostro Stato, ma invece valorizzare oggi il settore pubblico attraverso la competizione dei privati che entrano insieme con il pubblico all'interno della pubblica amministrazione, e soprattutto nell'economia. Pertanto, signor Ministro, quello che noi le chiediamo come Gruppo parlamentare Forza Italia è

le confermo innanzitutto che il Governo intende, conformemente a quanto previsto dal DEF, procedere all'operazione di dismissione e razionalizzazione del patrimonio dello Stato e delle sue partecipazioni per un ammontare complessivo di 20 miliardi nel triennio pari all'1 per cento del PIL. Lei ha opportunamente ricordato che questo tipo di operazione non è semplicemente volta a contribuire alla riduzione del debito pubblico, perché tali risorse a questo saranno orientate per legge. anche e soprattutto a portare in un'azione politica industriale maggiore efficienza in diversi settori che, in qualche caso, sono gestiti in modo efficiente efficiente ed efficace da parte della pubblica amministrazione; in qualche altro caso sicuramente il contributo alla gestione privatista potrà portare dei benefici. Per fare questo, per azionare questa politica di sviluppo industriale, serve come presupposto una buona reputazione. Ed è quello che questo Governo sta in qualche modo costruendo e che ha trovato sostanza nella buona risposta per quanto riguarda il collocamento dei BTP valore e nell'attenzione da parte dei soggetti finanziatori, anche internazionali. Con questi presupposti e con questa fiducia costruita grazie all'azione del Governo ultimi mesi - ringrazio il Parlamento per aver supportato questo tipo di politica - possiamo affrontare il programma di privatizzazioni e di razionalizzazioni. Ribadisco - come ho fatto in altra sede - che questo programma non prevede la cessione del controllo, che verrà comunque garantito. Per quanto concerne la cessione di immobili non funzionali all'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche, ricordo che, che, con il decreto-legge n. 75 del 2023, in particolare l'articolo 28-*quinquies*, proprio presso il Ministero dell'economia e delle finanze abbiamo istituito una cabina di regia con funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, che - come il senatore sa - è diffuso in molte agenzie, enti e settori e necessita

dei nostri BTP, che sono andate "a ruba" proprio nei mesi scorsi. Questo a dimostrazione di come si stia facendo oggi una politica economica che viene vista con grande interesse anche dagli investitori esterni. Bene quindi avviare questo piano. Noi, come Forza Italia, da tempo stiamo puntando a un'azione di questo genere, che - come dicevamo - non è un'azione di dismissione; non dobbiamo vendere i gioielli di Stato, ma dobbiamo efficientare sempre meglio e di più i servizi pubblici. Lo sta facendo Forza Italia, con il suo segretario Antonio Tajani. È grazie anche a questo che abbiamo accolto nella Nota di aggiornamento al DEF questa proposta, che vale vale 20 miliardi di risparmi in tre anni, che, anche alla luce di quelli che saranno prossimamente i vincoli europei e i nuovi approcci che dovremo avere con il Patto di stabilità, sono certamente risorse che si liberano per poter fare altro. Ministro, attendiamo l'evoluzione sicuramente in positivo di questo

(SVP-PATT, Cb))*. Signor Ministro, sono consapevole che lei ha ben altri problemi da risolvere che non questo. Però, purtroppo, qui il problema nasce da una circolare del suo Ministero e io dovevo rivolgermi a lei. Si tratta di questo: come sappiamo, gli impianti di produzione di energia eolica e solare fotovoltaica necessitano di condutture che di solito sono sotterranee e portano la corrente elettrica dal luogo di produzione alla centrale di distribuzione. Della centrale di distribuzione in poi è responsabile l'azienda che si occupa della fornitura dell'energia elettrica ai diversi utenti, mentre prima è responsabile l'azienda che produce l'energia elettrica. È evidente che quelle condutture, seppur nel sottosuolo, costituiscono una limitazione delle possibilità e delle potenzialità d'uso del territorio da parte della comunità che vive nel Comune di riferimento. È previsto un indennizzo, è previsto che venga dato qualcosa in cambio di un tale impatto: ai sensi della circolare del suo Ministero, si tratta di 800 euro fissi all'anno, a prescindere dalla quantità degli impianti presenti. Quindi, se in un Comune ci sono 200 pale eoliche e in un altro ce n'è una sola, sempre 800 sono gli euro; dove scorrono sotto terra decine di chilometri di cavi e dove scorrono 20 metri, è uguale. Io credo che ci sia un'evidente sperequazione rispetto a enti locali che

al canone unico patrimoniale dovuto per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuata, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, è stata oggetto di una norma di interpretazione autentica con il decreto-legge n. 146 del 2021, che ne ha chiarito la portata. Tale norma di interpretazione costituisce un presidio a tutela degli utenti finali del servizio, che diversamente si sarebbero visti gravati, per effetto del cosiddetto fenomeno della traslazione, del maggior onere sopportato dalle aziende erogatrici, con il conseguente aumento delle tariffe del canone unico patrimoniale applicabili alle occupazioni permanenti del territorio comunale. Detto ciò, è chiaro che il Parlamento si

parlamentari, di modificare o integrare questo tipo di interpretazione che, nel 2021, in qualche modo ha circoscritto e ha definito il tipo di contributo dovuto.

Meloni da lei predisposta avete introdotto la *top ten* delle nuove tasse. Avete aumentato l'IVA sui prodotti per la prima infanzia; l'IVA sui prodotti intimi femminili; le tasse sui tabacchi da inalazione; le tasse sui liquidi delle sigarette elettroniche; la cedolare sugli affitti brevi. Ancora, avete aumentato le tasse sulle plusvalenze sugli immobili ristrutturati; le ritenute sui bonifici edilizi; le ritenute sui professionisti per gli interventi edilizi; le tasse su immobili all'estero infine, le tasse sui lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, introducendo una nuova fattispecie di tassazione. Ora, al di fuori di questa *top ten*, arriva la questione delle ultime ore. Avete eliminato anche l'esenzione sull'Irpef agricola, che che valeva 248 milioni a favore degli imprenditori agricoli, introdotta nel 2015 dal Governo Renzi e dal ministro Martina. Noi le vogliamo chiedere: ma almeno una tassa riuscite a toglierla mentre ne introducete altre dieci? Ci può dire qualcosa

soluzione di cui si sente parlare in queste ore, infatti, è di fatto una presa in giro. È una soluzione a costo zero ed è una soluzione che si applicherebbe su una fascia, che andrebbe comunque già in esenzione. Insomma, provate per una volta a togliere una tassa, anziché introdurne

di dire, o si è dimenticato di citare quei pochi, miseri 16 miliardi di tasse in meno che questo Governo ha in qualche modo sgravato ai cittadini italiani più bisognosi Al netto di questo, il tema dell'Irpef agricola è già stato posto al presidente Meloni proprio ieri alla Camera dei deputati, in sede di *question time*. Voglio semplicemente dire che cercato, nella nostra politica di bilancio, in una situazione di generale incertezza geopolitica, una una serie di misure selettive a favore in particolare delle categorie e dei settori più colpiti dalla situazione di crisi internazionale e anche con riferimento agli imprenditori agricoli, quelli provati dalla siccità, dalle fitopatie e dalle tante emergenze manifestatesi nell'ultimo anno. A tal fine, ricordo che l'ultima legge di bilancio ha destinato 300 milioni di euro al nuovo fondo emergenza, sia per interventi a sostegno del comparto agricolo, sia per la pesca e la acquacoltura. nel finanziare il fondo indigenti, si sono tutelate le filiere italiane a vantaggio dei nostri agricoltori e di tutto l'indotto agroalimentare. Infine, sono stati apportato correttivi alla legge n. 102 del 2004 in relazione alla disciplina dello stato di calamità e della sospensione delle rate dei mutui. Tali misure, orientate a specifiche categorie, hanno sostituito i precedenti interventi di carattere generalizzato. Fermi restando quindi gli interventi già adottati e in precedenza ricordati, nonché tutte le altre misure agevolative vigenti per il comparto agricolo, è in corso di valutazione l'intervento in materia di esenzione dall'Irpef per gli imprenditori agricoli che necessitano di un effettivo sostegno, eventualmente prevedendo specifiche franchigie. Tale misura, quindi, potrà essere inserita nel primo veicolo normativo utile, che potrebbe essere anche il decreto-legge milleproroghe, attualmente all'esame della Camera dei deputati. *(Applausi)*.

ci ha confermato che effettivamente il tema dell'aumento dell'Irpef c'è stato eccome. Noi abbiamo vissuto nella paradossale situazione nella quale, quando i trattori e le proteste degli agricoltori sono iniziate, quasi quasi questo Governo cercava di negare il fatto di aver aumentato le tasse a quella categoria. Poi, come sempre, la realtà prende il sopravvento sull'immaginazione e anche sul fatto che si sposti il problema verso l'Europa, che ovviamente ha le sue responsabilità, ma non ha la responsabilità - come in questo caso denunciata da Italia Viva come primo partito - di aver aumentato le tasse agli agricoltori, quando - e lo ricordo - il Governo Renzi le ha diminuite. Questa è la verità. Oggi il ministro Giorgetti ci dice che forse nel milleproroghe, attraverso il meccanismo delle franchigie, verranno diminuite queste tasse. con grande franchezza che mi sarei aspettata altro da lei oggi, signor Ministro; tanto più che voi avete preso più volte la parola sui giornali per dire che era un'ingiustizia la cosa che voi stessi avete fatto dentro quel Governo. Non potete fare la politica dei due forni: in Consiglio dei ministri votate l'aumento delle tasse e sui giornali invece dite ai cittadini che voi le vorreste diminuire. *(Applausi)*. Non funziona più. Volete fare qualcosa di serio? Mettete mano davvero alle risorse del Paese, perché nelle cose che avete voluto fare, comprese numerose marchette, siete stati particolarmente efficaci. Allora, cercate di dare una mano agli agricoltori, diminuite le tasse, ripristinate le misure come aveva fatto il Governo Renzi. Dimostrate di essere seri in questo Paese e non attaccati solo ed esclusivamente alla propaganda, perché la propaganda si sta smantellando da sola. La verità sta prendendo il sopravvento sul vostro racconto e sull'immaginazione. E quei trattori vi stanno dicendo che è facile dire di stare dalla parte del popolo, quando poi bisogna governare e dimostrare di essere davvero dalla parte dell'economia italiana, dell'agricoltura italiana, dell'*export* italiano e di chi ogni giorno fa una discreta fatica per cercare di arrivare alla fine del mese.

dato il recente affidamento della Società infrastrutture Milano-Cortina a favore dell'impresa Pizzarotti, per un progetto *light* di 81,6 milioni e il non meglio precisato extrabudget di cui non si conoscono i costi e i dettagli. Preciso che il termine extrabudget è stato indicato il 30 gennaio 2024 nel comunicato stampa della Fondazione Milano-Cortina «per la realizzazione di alcuni allestimenti, ad oggi non previsti per lo svolgimento delle gare». Riassumendo l'*iter* travagliato per quest'opera, ricordo che in data 11 gennaio 2019 è stato ufficializzato il *dossier* della candidatura italiana alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026,

purtroppo solo con la pubblicazione del bilancio consuntivo. Apprendiamo inoltre dai documenti di gara che parti consistenti di forniture essenziali alla funzionalità della pista sono state trasferite a carico della stazione appaltante e che sono indicati 3.925.000 euro di lavori in amministrazione diretta, come i costi reali del taglio del pregiato lariceto di bassa quota, esteso su oltre 5 ettari. Tutto ciò premesso, si chiede di sapere se il signor Ministro sia a conoscenza dell'ammontare dei reali costi annuali della futura gestione dell'impianto e quando intenda rendere pubblica l'eventuale documentazione; su quali enti ricadranno le spese di gestione della pista e quali sono gli accordi istituzionali in essere per garantire la sostenibilità economica futura dell'impianto; quali sono i costi sostenuti fino ad oggi dalle diverse pubbliche amministrazioni, dal Comune di Cortina, dalla Regione Veneto, dallo Stato italiano, in particolare nel sostenere gli studi di sostenibilità economica dell'opera e delle diverse consulenze, i diversi progetti che sono stati affrontati e abbandonati, i costi di demolizione della vecchia pista, la messa in sicurezza del territorio.

ricordo che nel piano complessivo delle opere olimpiche di cui al DPCM 8 settembre 2023 è incluso l'intervento Cortina sliding center (lotto 2) di riqualificazione della pista Eugenio Monti, destinato alla rigenerazione delle aree contermini, all'adeguamento della viabilità e alla realizzazione di nuovi spazi e percorsi per la valorizzazione delle qualità identitarie. Per l'intervento è previsto un costo totale di 118,424 milioni di euro, di cui 81,6 per per la realizzazione delle opere. La copertura di tali oneri è, per la quota di 117,484 milioni di euro, a carico di risorse statali e, per 470.000 euro, a carico del Comune di Cortina d'Ampezzo e della Provincia di Belluno, per ciascun ente. Tali risorse sono state ritenute sufficienti in fase di razionalizzazione progettuale; fase nella quale sono state ridotte tutte le infrastrutture fisse non necessarie all'utilizzo della pista nel periodo successivo ai giochi olimpici, riducendone il costo di costruzione, l'impatto sul territorio e il costo di gestione. Per quanto riguarda la richiesta inerente alla futura sostenibilità economica dell'impianto, il cosiddetto piano di *legacy*, ricordo che già in fase di candidatura la Regione Veneto, il Comune di Cortina d'Ampezzo e le Province autonome di Trento di Bolzano hanno sottoscritto, in data 29 marzo 2019, una lettera di intenti. Da ultimo, il Comune di Cortina d'Ampezzo, con la deliberazione n. 13 del 18 gennaio 2024, ha formalmente identificato gli *asset* sui quali costruire il piano di *legacy* richiesto e ha individuato nella Seam Srl il veicolo societario gestore del relativo piano. Entrando nello specifico, sulla base delle informazioni fornite, risulta che tale appalto sia stato aggiudicato sulla base di un computo metrico che considera le opere da realizzare e che, con un riferimento ai costi di demolizione della vecchia pista, il consuntivo del quadro economico dell'intervento riporta un importo di 2.829.564 euro, a fronte di un importo finanziato di 3.812.700 euro, del Consiglio dei ministri dell'8 settembre 2022. Infine, con riferimento alla richiesta di costi complessivamente sostenuti fino ad oggi da diverse pubbliche amministrazioni per il progetto di riqualificazione della pista Eugenio Monti, sulla base dei dati forniti dal commissario straordinario, il dato relativo della spesa complessiva sostenuta ammonta a 6.110.905,76 euro. Tale spesa ricomprende, oltre all'importo precedentemente indicato di 2.000.829.564 euro per la demolizione della vecchia pista, tutti i costi sostenuti per studi, rilievi, sondaggi, indagini, servizi tecnici, progettazione, verifica e progettazione, pratiche amministrative, monitoraggio e spostamento dei sottoservizi.

lei stesso ha dichiarato che sta cominciando a pentirsi di queste Olimpiadi, salvo poi ritrattare e dire che è stata una battuta. A me sembra che a questo proposito non si possano fare delle battute, perché la realizzazione della pista da bob è un affare serio, che sta facendo fare una

per il futuro sul territorio e sulle future generazioni. Non c'è niente da fare, non sentite ragione, non si riesce a mettere la retromarcia su questa opera

un progetto *light,* ma poi ci saranno opere accessorie con un extrabudget*,* perché non si può fare una figuraccia in mondovisione con una pista ridicola richiesta dal ministro Salvini. È chiaro che avremo bisogno dell'impianto di illuminazione all'interno e all'esterno,

il 7 agosto 2023 il Governo italiano ha presentato alla Commissione europea la rimodulazione complessiva del PNRR con l'inserimento del capitolo REPower EU e, proprio al fine di rinvenire le risorse per finanziare i nuovi investimenti del citato piano, ha proposto il definanziamento dal PNRR di investimenti per un importo pari a 15,9 miliardi.

il nuovo decreto-legge che punta proprio a garantire la copertura finanziaria di questi investimenti, soprattutto comunali, usciti dal PNRR e che il provvedimento all'esame ha anche l'ambizioso compito di trovare i fondi per accompagnare tutte le nuove misure inserite nel PNRR.

oltre che nella dimensione del provvedimento, proprio nella gestione dei 21,4 miliardi rimodulati che servono per la revisione del Piano e soprattutto nella difficoltà di dettagliare i fondi sostitutivi per circa 13 miliardi di progetti definanziati dal nuovo PNRR.

si apprende, sempre da organi di stampa, che ci sia un certo disaccordo o disappunto. Entrambi i fondi sono utilizzabili, sì, ma con forti limitazioni, infatti il primo ha creato obbligazioni giuridicamente vincolanti e quindi difficili da definanziare, il secondo, com'è noto, ha un vincolo di destinazione con l'80 per cento nelle Regioni del Mezzogiorno ed è evidente quindi che è davvero necessario conoscere qui in Parlamento il quadro aggiornato degli interventi ricompresi. Lo abbiamo più volte chiesto, già con l'affare assegnato nelle Commissioni 4a e 5a. Pertanto, le chiediamo, Ministro, in che modo si intenda sopperire alla carenza di liquidità causata dai ritardi della liquidazione delle rate e dalla rimodulazione al ribasso degli importi e quali saranno le fonti di finanziamento delle opere comunali prima inserite e poi espunte dal PNRR. Inoltre, chiediamo di sapere qual è la tempistica per l'adozione del decreto PNRR-*quater*, quali risorse sono previste previste a copertura dello stesso e qual è lo stato d'avanzamento delle misure e degli interventi ricompresi nel Piano nazionale complementare. *ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, in relazione al primo quesito posto, ricordo che per gli interventi finanziati nell'ambito del PNRR la liquidità è assicurata dal sistema di norme vigenti attraverso l'istituto delle anticipazioni. sono infatti resi disponibili per gli interventi da realizzare anticipi nella misura del 10 per cento, percentuale rilevabile su motivata richiesta delle amministrazioni titolari degli interventi. Tale meccanismo non subisce modifiche per effetto della rimodulazione del PNRR concordata in sede europea. Per quanto attiene alle fonti di finanziamento delle opere comunali non più incluse nel PNRR, si evidenzia che relativamente agli interventi già finanziati a valere sulle risorse dell'articolo 1, comma 139, della legge n. 145 del 2018, cosiddette medie opere,

a essere finanziati a valere sulle risorse recate da tali autorizzazioni di spesa, senza alcuna conseguenza dovuta all'uscita dal PNRR, dovuta - lo ricordo fatto che buona parte di queste opere per le loro caratteristiche purtroppo non potevano nel PNRR essere finanziate. Per gli altri interventi di competenza dei Comuni in parte usciti dal PNRR, quali i piani urbani integrati, sono in corso gli approfondimenti per l'individuazione delle risorse necessarie ad assicurarne la continuità. Relativamente all'adozione del decreto-legge PNRR cosiddetto provvedimento necessario per dare corso ad alcune delle nuove misure previste dal Piano, comunico che il testo è in fase di elaborazione e sarà sottoposto a breve al Consiglio dei ministri. Per quanto riguarda lo stato di avanzamento del Piano nazionale complementare, sulla base delle comunicazioni delle amministrazioni titolari e delle risultanze del sistema di monitoraggio, è in corso di predisposizione l'aggiornamento del *report* periodico sullo stato di avanzamento degli interventi che, come i precedenti, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato.

del PNRR e non del 10 per cento degli anticipi che, sì, vengono dati ai Comuni; al di là di questo, rimane però il fatto che abbiamo comunque l'assenza di dati certi sullo stato d'avanzamento delle misure e degli interventi ricompresi nel Piano nazionale complementare e la conseguente assenza di garanzia per gli enti locali, perché alcuni di tali continuano a portare avanti i progetti, nonostante da parte del Ministero dell'economia e delle finanze alcune risorse non siano state ancora erogate, proprio in virtù di capire quali finanziamenti rimarranno

di concentrare l'80 per cento delle misure nelle Regioni del Mezzogiorno. In attesa di leggere il decreto PNRR-*quater*, pertanto, la nostra allerta resta massima, sperando che non vengano tradite le aspettative degli amministratori locali.

nella legge di bilancio per il 2024 è stato previsto di escludere dal calcolo dell'ISEE il patrimonio detenuto in titoli di Stato, fino a un limite di 50.000 euro che in precedenza rientrava nel calcolo. Lo scorso anno abbiamo avuto un successo notevole nella vendita di titoli di Stato (32 miliardi nelle emissioni di giugno e di ottobre). È chiaro che questa misura incentiverà ulteriormente l'acquisto di titoli di Stato Tuttavia, l'INPS ha chiarito che la misura, per entrare in vigore, ha necessità di una modifica un regolamentare, quindi, ad ora, abbiamo ancora il regime precedente. Le chiediamo quindi quali sono le iniziative, sue e del Ministero, per arrivare a un'effettiva attuazione di questa misura con la modifica del regolamento.

dicembre 2023, n. 213, all'articolo 1, comma 183, ha previsto l'esclusione dal calcolo dell'ISEE, fino a un valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. Appena entrata in vigore la disposizione, sono state svolte riunioni tecniche al fine di individuare il perimetro dei suddetti prodotti finanziari e titoli di Stato ai quali applicare l'esclusione dal calcolo dell'ISEE. In particolare, si tratta di titoli di Stato, buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato, libretti di risparmio postale e altri prodotti finanziari con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. La notizia positiva è che lo schema di decreto è già stato trasmesso dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale ha concluso le attività istruttorie di competenza e trasmetterà molto presto lo schema, per il completamento del suo *iter*, al Consiglio di Stato per l'acquisizione del parere,

cui sarà completato, sarà infatti possibile per tutti i cittadini italiani aggiornare il proprio ISEE e, in prospettiva, avere maggiori garanzie anche rispetto alle decisioni di investimento prossime venture e per quanto riguarda i loro risparmi.

dà notizia che ormai, a breve, questa misura diventerà operativa. Ciò è molto importante anche perché la quota di titoli di Stato di debito pubblico detenuta dagli italiani

anche in seguito alla stretta, che era sacrosanta, della misura del reddito di cittadinanza. La ringrazio, signor Ministro, e le auguriamo di proseguire in questo ottimo lavoro.

questo programma, che peraltro va controcorrente rispetto a una fase in cui tutti i grandi Paesi avanzati registrano un rinnovato protagonismo diretto dello Stato nelle politiche di sostegno del sistema industriale. Il ministro Giorgetti, che saluto, ha dichiarato che le dismissioni sono tra i principali strumenti per abbattere il debito pubblico nella manovra triennale. Eppure 20 miliardi, l'obiettivo del programma, sono solo lo 0,7 per cento dello *stock* di debito delle PA. Privatizzare peraltro vuol dire rischiare di rinunciare a dividendi che in non pochi casi rischiano di essere superiori rispetto al risparmio in termini di minori interessi sul debito. La presidente Meloni il 12 dicembre ha affermato che le privatizzazioni non diventeranno mai svendite. Vorrei ricordare al signor Ministro che il 20 novembre il MEF ha ceduto il 25 per cento di MPS a 2,92 euro per azione, incassando 920 milioni. ci obbligava a fare quell'operazione in quel momento. Da allora, il valore del titolo è progressivamente aumentato e oggi la quotazione è pari a 3,57 euro, cento in più. Se avessimo fatto oggi questa operazione e non il 20 novembre, avremmo incassato 200 milioni di euro in più lo sottolineo. Non bisognava essere scienziati per sapere che in una fase in cui tutte le banche stanno aumentando i propri margini di redditività, i corsi sarebbero saliti. Ad oggi, Presidente, abbiamo informazioni frammentarie su quali società saranno interessate dal piano. Si è parlato in particolare di Poste e Ferrovie dello Stato. Sono ipotesi che ci preoccupano e ci vedono molto critici per la valenza di queste società, ma anche per il mercato in cui operano, che vede un grande attivismo e un grande peso di soggetti come Amazon e MSC. La logistica è un mercato particolare e noi rischiamo di privatizzare in questo contesto società di grande rilevanza. Allora, Presidente, chiediamo di sapere una volta per tutte le linee di indirizzo di questo programma, le società coinvolte, le motivazioni industriali e non solo finanziarie, le tempistiche, le modalità di esecuzione e l'impatto finanziario, non solo le previsioni di ricavo, ma anche a quanti dividendi a quanti dividendi andremo a rinunciare, privatizzando parti delle società partecipate. Chiediamo insomma di sapere i contorni e gli obiettivi, al di là delle poche dichiarazioni frammentarie, di un programma di privatizzazioni che giudichiamo molto negativamente, perché incentrato solo su logiche di cassa, senza un chiaro disegno di politica industriale, che riteniamo nel complesso contrario agli interessi del Paese.

Misiani, nessuno di noi si ritiene uno scienziato. Al MEF ci sono dei poveri politici, che parlano con la gente e cercano non di annullare un debito pubblico che hanno ereditato, ma di gestirlo al meglio, cercando di aumentare la credibilità e la reputazione del Paese e di convincere i risparmiatori internazionali e nazionali a sottoscrivere e a rinnovare la loro fiducia nei confronti del Paese. Questo è avvenuto in modo sorprendente, soprattutto per quegli scienziati che annunciavano il disastro quando questo Governo è entrato in carica. *(Applausi)*. Detto questo, contesto la sua affermazione che in giro per l'Europa fanno esattamente il contrario di quello che sta facendo il Governo italiano. La cassa depositi e prestiti tedesca proprio in settimana ha "privatizzato" una parte di Deutsche Post, esattamente quello che intende fare il Governo italiano, ma il programma del Governo italiano non è volto semplicemente ad abbattere il debito pubblico, perché siamo assolutamente consapevoli che ciò non può avvenire per questa via. È un processo che - come

che si è allargata in settori come quelli delle banche e delle assicurazioni e ha permesso a Poste di sopravvivere in condizioni di economicità e di efficienza.

ma anche il processo di privatizzazione sarà orientato in qualche modo a privilegiare i risparmiatori italiani e i dipendenti, a cui crediamo sia giusto riconoscere la possibilità di aderire in forma preventiva e prioritaria. Nel ribadire che non prevediamo di cederne il controllo, ci muoveremo sempre nella logica della difesa dell'interesse generale. di riferimento relativi al momento in cui allocare o non allocare dipendono anche da una serie di circostanze, tutte tese a rafforzare la credibilità del Paese, anche, se vogliamo, in determinate fasi e congiunture.

la valutazione di quando procedere e di quando non procedere sarà soggetta a valutazioni di diverso tipo e di interesse generale, non lo faremo semplicemente perché non siamo in grado di finanziare le casse dello Stato (abbiamo infatti dimostrato, con tutte le emissioni di titoli del debito pubblico, di essere in grado di farlo in ogni situazione), ma semplicemente perché questo tipo di politica sia corretta in termini di politica industriale. Concludo dicendo che è vero che in qualche caso privatizziamo. In qualche caso, però, siamo chiamati

gli chiediamo di rassicurare anche i cittadini italiani, i lavoratori e le lavoratrici di quelle imprese e tutti gli *stakeholder*. È tempo che il Governo venga in Parlamento, il luogo della democrazia, a spiegare le ragioni del piano e le motivazioni di politica industriale di ciascuna operazione che verrà messa in campo, e non soltanto gli obiettivi di incasso per tentare di tenere su un sentiero discendente il rapporto debito-PIL. Questa, infatti, è la vera motivazione del piano. spiegare, lo ripeto, a quanti dividendi andiamo a rinunciare, perché il rischio che intravediamo è che si rinunci a dividendi superiori rispetto a quello che si andrebbe a risparmiare in termini di minori interessi sul debito pubblico. Se le cose stanno nei termini della risposta del Ministro, purtroppo rimaniamo convinti che l'unica vera motivazione di questo piano sia fare cassa. Attenzione, sì, facendo cassa, ma rischiate di farla a caro prezzo per il Paese, rischiando di privatizzare società che stanno ricevendo e riceveranno miliardi di euro del PNRR, risorse pubbliche che aumenteranno, presumibilmente, il valore di queste società strategiche per il Paese. Allora, che ci sia il rischio di una svendita di *asset* strategici di grande valore e di grande redditività per le casse pubbliche, per lo Stato e per i cittadini contribuenti è un rischio concreto e purtroppo le parole del Ministro non ci hanno rassicurato sotto questo e altri profili.